Onorevoli colleghi, duecento anni fa, il 25 maggio del 1810, un gruppo di patrioti proclamò a Buenos Aires la Giunta governativa provvisoria del Rio de la Plata. Fu questa «Rivoluzione di maggio» il battesimo della Nazione argentina. Di questo manipolo di padri fondatori delle libere istituzioni argentine faceva parte il nostro compatriota generale Belgrano, il quale, formatosi alla scuola di Galiani e di Genovesi, non solo combatté con il braccio e con la mente per la libertà e l'indipendenza del Paese che aveva accolto la sua famiglia, ma si preoccupò del suo avvenire, fondando scuole e istituti di cultura, fornendo un contributo decisivo politico e intellettuale all'apertura dei mercati e dell'economia che resero prospera l'Argentina. Di questa prosperità, con orgoglio, voglio ricordare oggi il contributo italiano. Quei milioni di emigranti che dalla prima metà dell'800, dopo la sconfitta del dittatore Rosas, anche all'eroismo di Garibaldi e dei suoi legionari, contribuirono alla grande stagione di progresso civile e sociale che si sviluppò sotto la Costituzione del 1853. Con questi sentimenti, dunque, di fratellanza e di profonda amicizia credo di interpretare il sentimento di voi tutti nel formulare alle autorità argentine gli auguri più sentiti per questo anniversario. Da quest'Aula del Parlamento, nel segno di quella bandiera che dopo aver sventolato a Milano nelle Cinque giornate attraversò l'oceano con la legione garibaldina, bagnata del sangue del patriota Virginio Bianchi e custodita a Buenos Aires come preziosa reliquia, vada alla Nazione argentina il saluto del Senato italiano e l'omaggio a quella bandiera bianca e azzurra che l'italiano Belgrano volle dare all'Argentina, a testimonianza indissolubile del legame che ha stretto e stringe ancor più oggi le nostre due Nazioni. Un saluto, inoltre, che vuole interpretare il sentimento di un popolo amico e delle centinaia di migliaia di connazionali che vivono in Argentina e lavorano con impegno per il suo benessere. La consapevolezza di questo contributo essenziale, delle comuni radici, ci spinga oggi a rafforzare il legame tra i nostri due Paesi, coinvolgendo a pieno i nostri giovani per riscoprire le ragioni dell'affinità profonda che ci lega.

con questa significativa celebrazione del 200° anniversario dell'indipendenza argentina. Lo dobbiamo alle centinaia di migliaia di nostri connazionali che vivono e operano in quel Paese: si tratta della più numerosa comunità italiana all'estero. Lo dobbiamo poi a quei milioni di nostri connazionali che con grandi sacrifici attraversarono l'oceano per dare un contributo decisivo alla costruzione e alla prosperità di quello straordinario Paese di cui oggi celebriamo l'indipendenza. Come ha ricordato lei, signor Presidente, l'indipendenza dalla dominazione straniera fu una battaglia combattuta in Argentina come in Italia in nome dei diritti della libertà e della costruzione di libere istituzioni rappresentative. È dunque particolarmente significativo che da quest'Aula parta oggi un messaggio alla Nazione argentina che rivolgo in particolare all'ambasciatore, signora Norma Nascimbene de Dumont, che assiste ai nostri lavori.

Credo, signor Presidente, che questa occasione importante debba essere di stimolo per rafforzare i rapporti fra i nostri due Paesi. Se siamo orgogliosi delle realizzazioni delle realizzazioni della collettività italiana, al cui servizio opera la più importante rete consolare di cui l'Italia dispone nel mondo, dobbiamo tuttavia essere consapevoli della necessità di andare oltre. La cultura italiana, per le ragioni che ha ricordato lei, signor Presidente, è un elemento costitutivo della Nazione argentina. Questo deve essere è elemento che deve spingere la nostra rappresentanza diplomatica, la nostra rete consolare e più in generale tutta la presenza italiana in Argentina ad andare oltre i pur fondamentali rapporti con la nostra collettività. Ci dobbiamo rivolgere al popolo argentino nella sua complessità e in particolare ai giovani e alle forze più dinamiche e produttive. Oggi, di fronte a una crisi che tanto duramente sta colpendo il nostro Paese e più in generale il nostro continente, dobbiamo essere consapevoli della straordinaria risorsa che rappresenta per noi questo storico e forte rapporto con un Paese che ha un'economia vitale. Dobbiamo essere consapevoli di quale straordinaria risorsa sia il rapporto che, grazie alla grande storia della nostra emigrazione, abbiamo con un continente - il Sud-America il cui sviluppo impetuoso apre oggi più che mai nuove e inedite possibilità alle nostre imprese e alle energie migliori del nostro Paese. Con questi sentimenti, a nome della Commissione affari esteri del Senato, mi associo quindi all'indirizzo di auguri alla Nazione argentina con cui lei, signor Presidente, ha aperto i lavori della nostra Assemblea. *(Applausi. CARLINO *(IdV)*. Onorevoli colleghi, signor Presidente, il 2010 è l'anno nel quale ricorre il bicentenario dell'indipendenza non solo dell'Argentina, ma di tutto un intero continente: duecento anni fa, infatti fu l'America latina intera che avviò un processo che avrebbe portato alla libertà del suo popolo. Il 19 aprile del 1810 fu cacciato infatti il governatore spagnolo dal Venezuela, il 20 luglio è stata segnata l'indipendenza della Colombia, il 16 settembre iniziò il processo di liberazione dal giogo spagnolo in Messico, e il 18 settembre è la ricorrenza dell'insediamento della prima giunta di Governo in Cile. oggi, 25 maggio, ebbe luogo la «Rivoluzione di maggio» argentina, che fu il risultato della rottura dei legami coloniali con la Spagna nel 1810, rottura che iniziò il percorso verso l'indipendenza, che finalmente ebbe luogo il 9 luglio 1816. Non possiamo pertanto ricordare l'indipendenza dell'Argentina senza inquadrare il movimento di liberazione in un contesto macroregionale, quando, dopo la barbarie del colonialismo, i popoli riuscirono ad affermare l'aspirazione dell'autodeterminazione, il principio che oggi costituisce la base del diritto internazionale su cui vigila l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il «fardello dell'uomo bianco», che si realizzò in un sistema imperniato su stermini di massa, sfruttamento schiavistico e ideologia razzista, ha scritto nel continente latino americano una delle peggiori pagine. Ed ancora oggi, sebbene l'Italia non abbia mai partecipato direttamente alla colonializzazione dell'area, credo che, come nazione europea, non possiamo ricordare l'indipendenza del continente latino-americano, senza premettere alla riflessione politica sull'oggi un *mea culpa* sui misfatti di ieri. Così come ha fatto Giovanni Paolo II il 12 ottobre 1992, nell'ambito della commemorazione del V Centenario dell'inizio dell'evangelizzazione del Nuovo Mondo, quando ha dedicato un pensiero agli *indios*, che per la storia sono stati i «figli di un Dio minore», affermando che «dobbiamo riconoscere in tutta sincerità gli abusi commessi, dovuti alla mancanza d'amore da parte di quelle persone che non seppero vedere negli indigeni dei fratelli, figli dello stesso Dio Padre». Con questo, colleghi, voglio dire che oggi non è soltanto il bicentenario dell'indipendenza politica dell'Argentina, ma ricorre il primo passo con il quale si è iniziato un più alto percorso di giustizia internazionale, di libertà, di autogoverno e di democrazia. L'Argentina riveste per l'Italia un significato particolare, in quanto, data la forte componente di italiani emigrati, rappresenta un'appendice viva e pulsante del nostro Paese. Tra il 1876 e il 1976, l'Argentina da sola ha infatti accolto circa l'11,5 per cento degli italiani milioni di italiani sono entrati in quella Repubblica durante un secolo, ed oggi che il tasso di presenza italiana sul totale della popolazione straniera si è mantenuto su percentuali considerevoli (siamo al 20 la comunità italiana in Argentina costituisce la quarta per italiani residenti all'estero e la più numerosa fuori dal continente europeo. Gli italiani hanno avviato imprese, ne contiamo 1.317 attualmente, si sono impegnati nella vita politica del Paese (si pensi che sono 70 i deputati di origine italiana eletti alla Camera e 14 al Senato), e hanno contribuito allo sviluppo culturale e sociale dell'Argentina. Per questo è importante che il Senato abbia voluto dedicare un momento particolare per ricordare, oggi, la Rivoluzione di maggio, poiché sono tanti gli italiani che, pur essendosi fortemente integrati nel tessuto argentino, mantengono un legame particolarmente stretto con il nostro Paese. questa occasione deve servire anche per chiedere al nostro Governo un maggiore impulso per tutelare davvero i nostri connazionali che vivono oltreoceano. Non possiamo festeggiare il bicentenario dell'indipendenza, infatti, se non vi sarà un concreta indipendenza economica del paese latino-americano.

*(IdV)*. Stavo parlando dell'indipendenza economica. Nel 2001, infatti, a seguito di quattro anni consecutivi di recessione, è scoppiata violentissima la crisi economica, finanziaria, politica e sociale. Il Governo italiano ha fatto molto: si è deciso lo stanziamento di 75 milioni per il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Tuttavia, questo non basta: ancora oggi sono oltre 180.000 gli italiani risparmiatori che non hanno partecipato allo *swap* proposto dall'Argentina nel 2005, perché ritenuto inaccettabile, e che aspettano di essere ripagati dal Governo argentino. La somma totale che il Paese sudamericano doveva al momento della crisi agli investitori italiani superava i 4 miliardi dì dollari, e, secondo uno studio condotto dall'*American task force Argentina* al gennaio 2005, la bancarotta argentina costava agli investitori italiani circa 11,3 miliardi di dollari e ha provocato un minor gettito per l'erario quantificabile tra i 4,2 e i 4,3 miliardi di dollari. In un periodo tanto difficile per la nostra economia, come Italia dei Valori chiediamo pertanto al Governo di adoperarsi con qualsiasi mezzo per conseguire un accordo transattivo con il Governo argentino che possa ripagare i cittadini italiani delle perdite. Chiudo, colleghi, affermando che davvero il modo migliore per festeggiare l'indipendenza di un grande Paese come l'Argentina è quello di aumentare gli sforzi per sostenere gli italiani all'estero, per ripagare i risparmiatori italiani che hanno investito nei cosiddetti tango-*bond*, per riformare una rappresentanza che non funziona, per dare sviluppo agli istituti di cultura italiana e agli organi di informazione bilingue. Dobbiamo insomma attuare progetti concreti per far sì che quegli «argentini che di cognome fanno Rossi» abbiano dal nostro Paese l'assistenza che davvero meritano. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la commemorazione del bicentenario della Rivoluzione di maggio del 1810 rappresenta un'opportunità irripetibile per sospingere noi argentini a pensare e riflettere insieme sul nostro passato, presente e futuro. Il 2010 ci consente di fare un bilancio della nostra storia e di pianificare un domani migliore per discutere e stabilire mete, obiettivi, politiche e strategie per concertare e realizzare un progetto di Paese. Consentitemi, quindi, una piccola considerazione su questo processo indipendentista che ha coinvolto anche la comunità italiana, contribuendo così a modificare la fisionomia del Paese, partecipando a una crescita industriale, agricola, commerciale senza precedenti. E proprio nel 1853, quando fu proclamata la nuova Carta costituzionale, che istituì in Argentina una Confederazione di Stati, venne riconosciuta l'importanza dell'immigrazione. Ruolo fondamentale nella difesa dell'immigrazione lo ha avuto un italiano, il generale Bartolomé Mitre, considerato uno dei fondatori della Nazione argentina, che fece inserire nell'articolo 25 della Costituzione la tutela dell'immigrazione. Altri personaggi italiani hanno contribuito a formare la storia dell'Argentina. Come non parlare del generale e patriota Manuel Belgrano, considerato uno dei padri fondatori dell'Argentina e ideatore della bandiera argentina? E con particolare orgoglio vorrei ricordare che proprio nell'interno del primo Governo patrio argentino erano presenti quattro membri di origine italiana su un totale di nove. Non sono qui per fare un elenco di illustri personaggi italiani che si sono susseguiti nel corso dei secoli, ma per ricordare anche gli eventi che hanno caratterizzato drammaticamente la vita tutto il popolo argentino, come la dittatura militare, la guerra delle Malvine, l'atroce e tragica vicenda dei *desaparecidos* e, da ultimo, la crisi economica del 2001. Attualmente l'Argentina si trova di fronte a nuove sfide e, come duecento anni fa, abbiamo davanti a noi cambiamenti mondiali che vanno al di là della semplice teoria. Siamo certi che l'attuale dinamica globale geopolitica e geostrategica tende alla creazione di molteplici poli di potere e, per questa ragione, si deve dibattere su queste nuove realtà per far sì di poter partecipare nuovamente nello scenario mondiale. Il Bicentenario sarà quindi per noi un ponte per continuare ad approfondire il dibattito in tutto il Paese. Uno scambio che ci consenta di essere concordi nella linea da seguire per crescere insieme. Per concludere, vorrei ricordare come il contributo di valori morali, di lavoro e di cultura dato dagli italiani nell'edificazione della società argentina è stato e continua ad essere straordinario. Gli italiani hanno lasciato un segno indelebile in questo Paese, e l'italianità dell'Argentina costituisce una preziosa risorsa, da trasformare in collaborazioni concrete con l'Italia. È anche in questa nuova e stimolante dimensione che ora siamo pronti a dedicare tutto il nostro impegno per garantire che lo spirito della Costituzione risulti ulteriormente e significativamente potenziato. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che si adopereranno attivamente per mantenere vivi e intensificare gli stretti legami tra i nostri Paesi, promuovendo e partecipando alle iniziative che si svilupperanno in ogni campo con l'Italia. Signor Presidente, come da lei ricordato e come ricordato dal presidente Dini e dai colleghi senatori che mi hanno preceduto,

Questa ricorrenza riguarda Paesi come il Venezuela, la Colombia, il Messico, il Cile e, proprio oggi, il 25 maggio, l'Argentina. Come ha ricordato il nostro ministro Franco Frattini, la scelta dell'Italia di celebrare questa importante ricorrenza conferma la nostra costante attenzione nei confronti di una regione alla quale siamo uniti da profondi rapporti sia storici che umani. Per noi celebrare l'indipendenza dell'America latina significa ricordare le centinaia di migliaia di italiani tra i quali tantissimi, lo voglio ricordare con orgoglio, provenienti proprio dal mio Veneto - partiti appunto verso i Paesi del Sud America. la nostra è una doverosa attenzione verso l'America latina, che si fonda su vincoli di sangue, su valori comuni, comuni basi culturali e ovviamente anche su interessi economici. Il percorso che portò all'indipendenza dell'America latina parla per un certo verso italiano, essendo idealmente cominciato proprio qui a Roma il 15 agosto 1805 con il giuramento di Monte Sacro. La presenza italiana nei Paesi dell'America latina, iniziata verso gli anni '80 del 1800, raggiunse quote impressionanti: basti pensare che il 60 per cento degli emigrati veneti approdò proprio in questi Paesi. Ad incentivare l'emigrazione transoceanica sicuramente c'era la possibilità di avere un viaggio gratis e la promessa di un pezzo di terra in proprietà. Concludo ricordando che il nostro Paese avrà un ruolo attivo nelle celebrazioni dell'indipendenza di tutti i Paesi latino-americani: si terranno infatti in tutto il territorio una serie manifestazioni per riflettere sul ruolo degli italiani nella nascita e nel progresso progresso di quelle Nazioni, alcune delle quali saranno promosse anche dalla società «Dante Alighieri», dall'Istituto italo-latino americano e dai singoli istituti italiani di cultura all'estero. *(PD).* Signor Presidente, a me sembra che non ci sia nulla di formale nello spirito con cui noi oggi in Senato ricordiamo il bicentenario dell'Argentina. Il nostro animo muove da un rapporto di amicizia tra due Paesi che sono legati da relazioni intense che vanno molto al di là della pur importante alleanza di due Stati sovrani. Al cuore dei nostri rapporti c'è un legame profondo tra donne e uomini che da un paio di secoli, ben prima che nascesse l'Italia, con il loro lavoro e i loro sacrifici hanno costruito il proprio destino, amando con pari intensità la terra dove si sono stabiliti e quella da cui sono partiti. L'Argentina si è impastata con gli italiani, prendendone le virtù ed anche i vizi. Il nostro è stato un viaggio senza *conquistadores*: nessuno sottometteva l'altro, ma si andava realizzando quel meticciato che Carlos Fuentes segnala come la vera identità latino-americana. Un'invasione fatta di umanità e di lavoro, senza armi e senza eserciti. Milioni di donne e di uomini di prima, seconda, terza e persino quarta generazione. Persone che sono andate in Argentina per cercare fortuna, che portano un nome italiano ed hanno il passaporto italiano. Molti di loro parlano poco la lingua italiana, solo perché i loro padri parlavano veneto, siciliano, friulano o calabrese. Tornano in Italia quando possono ed hanno nostalgia per l'Italia. Ma sono leali e operosi cittadini argentini. Il 25 maggio non è solo una celebrazione perché, come tutte le storie, è fatta anche di ombre e di appannamento delle libertà: è successo in Italia con il fascismo e in Argentina con le dittature militari. In questo intreccio di sentimenti e di rimorsi, di nostalgie e di affetti, c'è la radice profonda del rapporto che lega l'Italia all'Argentina. E c'è anche la spiegazione dei tanti legami culturali, economici e politici che nell'800, nel '900 ed oggi rendono i due Paesi così affini e così intimamente vicini. Ad agosto, quando «La Scala» significativamente presenterà l'«Aida» di Giuseppe Verdi al Teatro «Colòn» di Buenos Aires, si potrà dire che un cerchio virtuoso si sarà chiuso. Ma al di là di questo specialissimo rapporto, insieme politico e sentimentale, sono numerose le ragioni per le quali il bicentenario interpella direttamente anche noi italiani e ci sollecita a riflettere non solo sull'amicizia tra i due Paesi, ma anche sull'Italia che abbiamo in mente. In primo luogo la storia dell'Argentina ci invita a non richiuderci a protezione dei nostri apparenti interessi, ma a ricercare con responsabilità una buona politica nazionale di accoglienza e integrazione. Per l'Argentina l'integrazione degli immigrati non è stata imposta dalle circostanze. È stata una precisa e lungimirante scelta politica che merita molto rispetto e molta considerazione. Negli ultimi cinquant'anni, e ancor prima col peronismo, l'altalenarsi dei cicli economici, anche molto gravi, ha determinato in Argentina un difficile succedersi di democrazia e di sonno della ragione. Molti esiliati politici argentini hanno trovato rifugio in Italia. Persone che non avevano alcuna intenzione di emigrare ma che, perseguitate, fuggivano dalla loro Patria. È da quel periodo tragico che nel nostro vocabolario è entrata una nuova e terribile, parola: *desaparecidos*. Quegli oltre trentamila giovani (un'intera classe dirigente) scomparsi nel nulla, buttati vivi dagli aerei, torturati e ammassati in fosse comuni, cercati dalle loro straordinarie "madri". E i figli di quei trentamila, fatti nascere dagli aguzzini per essere venduti o ceduti, cercati uno ad uno dalle loro eroiche "nonne", le *abuelas*. Estela Carlotto e Lita Boitano, due donne tenaci dal cognome italiano, sono diventate simbolo della lotta per la dignità; hanno vissuto nei processi in Italia contro gli aguzzini dei loro cari un riscatto ed una, parzialissima, pacificazione. Nel XXI secolo le cose sono cambiate, signor Presidente, ed oggi è l'Italia ad essere diventata terra d'immigrazione. Quell'Italia di cui ieri la Conferenza episcopale italiana ha denunciato il suicidio demografico. Un'immigrazione di cui noi abbiamo bisogno e che vogliamo legale. Il principio di legalità è condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente. Senza integrazione, anche l'immigrazione legale finisce fatalmente per diventare un pericoloso focolaio di squilibri sociali. C'è in Italia il dovuto rispetto ed amicizia nei confronti di chi, legalmente, viene da noi a lavorare? Ci sono le premesse politiche e culturali di una buona integrazione? Queste domande non dovremmo nemmeno porcele, ma siamo costretti a farlo sentendo un autorevole membro del Governo dichiarare con molta disinvoltura che «gli immigrati sono una risorsa negativa». La storia dell'Argentina, che nell'integrazione ha costruito la sua identità nazionale, ci indica qual è la qualità dell'accoglienza che il mondo si aspetta da noi. Rigorosi nel chiedere rispetto per le nostre leggi, ma leali nel dare il benvenuto a chi viene legalmente e ci porta il suo lavoro. Larga parte degli argentini ha almeno un nonno di origine italiana. Ne costituisce oggi testimonianza - è stato ricordato poco fa il cognome italiano di un terzo dei membri del Parlamento argentino. Signor Presidente, tra un secolo, ma forse molto prima, nel Parlamento italiano siederanno tanti i cui cognomi non saranno italiani, cognomi che riveleranno l'origine di tanti nuovi parlamentari, indicheranno da dove, da quale continente provengono. In quel momento il clima politico e la pace sociale del nostro Paese dipenderanno dallo spirito e dai modi della nostra attuale cultura di accoglienza. Se oggi seminiamo inimicizia e ostilità nei confronti degli immigrati, per domani non aspettiamoci nulla di diverso. La seconda questione per la quale la storia dell'Argentina ci riguarda ha a che fare con i progressi del processo di integrazione tra i Paesi del continente sudamericano. Anche le Nazioni del Sudamerica stanno capendo come nel mondo globale nessuno Stato possa farcela da solo. Traiamone una lezione per l'Italia. L'euro, la moneta unica che oggi è sotto attacco dalla speculazione, non basta più a proteggere l'Europa. Per salvare l'Europa è nostro dovere agire con forza nella direzione della sua integrazione politica. Nel mondo contemporaneo l'euro e la BCE sono l'unica moneta e l'unica Banca centrale a non avere dietro uno Stato, un'unica politica economica e fiscale, un unico impianto normativo di base. Presidente, ho finito. Cito solo la terza questione sulla quale il bicentenario dell'Argentina ci interpella e interpella il nostro Governo: essa riguarda la nostra abitudine di rendere opachi persino i più grandi appuntamenti della nostra storia. In questi tempi anche la democrazia argentina, come l'Italia, è terra di competizioni e di tensioni politiche. Ma in Argentina mai a qualcuno è venuto in mente di giocare politicamente con l'unità del Paese. Per questo da oggi, e per un intero anno, l'Argentina intera vivrà l'emozione di un grande Paese, felice d'essere libero e unito, da Buenos Aires alla Patagonia. Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ha indotto alcuni parlamentari italiani e, addirittura, alcuni membri del Governo, a definire «inutili e retoriche» le celebrazioni. Sono posizioni politiche che il Partito Democratico respinge. L'Unità d'Italia può essere celebrata degnamente solo proponendo al Paese politiche di unità e di condanna dei bassi istinti di divisione. Questo è lo spirito con cui da oggi l'Argentina celebra il suo bicentenario. Ma se questo spirito non fosse anche il nostro, se lasciassimo venir meno la tensione morale verso l'Unità d'Italia, anche questa nostra celebrazione per il bicentenario argentino si tingerebbero di retorica. Signor Presidente,

Caro Presidente, carissimi colleghi, in occasione del bicentenario dell'indipendenza argentina, siamo qui riuniti per celebrare con solennità questo importante evento storico che ha segnato la nascita della grande Nazione sudamericana. Infatti, la "Rivoluzione di maggio", che oggi in questa sede ricordiamo, fu il risultato della rottura, nel lontano 1810, del legame coloniale con la Spagna,

La "Rivoluzione di maggio" fu sì un processo storico ma anche un sogno divenuto realtà, dove uomini colti, come Mariano Moreno, Manuel Belgrano Juan José Castelli, rivendicarono il diritto ad essere sovrani. Ma perché questa sovranità diventasse effettiva, era necessario che altri valori come la libertà e l'uguaglianza fossero anche presenti. Credo, cari amici, che oggi dobbiamo commemorare il bicentenario partendo proprio da quei valori di sovranità, uguaglianza e libertà, cioè a dire la democrazia stessa come un compromesso permanente. Dal 1810 si è fatto molto per difendere questo sogno dei padri fondatori i festeggiamenti per il bicentenario devono servire perché la società argentina abbia una nozione più chiara della sua identità e ogni cittadino possa riconoscere in essa un senso di appartenenza che lo renda orgoglioso. Vorrei sottolineare che, grazie all'immigrazione italiana

perché gli italiani lavoravano la terra con le proprie mani, e un tempo ha avuto l'onore di occupare il settimo posto tra le Nazioni e, dopo la guerra, è stata solidale con l'Europa dando da mangiare a tanta gente. Con questo voglio dire grazie anche a voi tutti, colleghi senatori, di maggioranza e di opposizione, chiedendovi allo stesso tempo chi di voi non abbia un parente che ha vissuto o vive ancora in Argentina. Per questo motivo, carissima Italia, questo umile senatore italo-argentino, che è arrivato nel Senato della Repubblica italiana rappresentando 13 Paesi dell'America latina,

È altamente probabile che sul calendario, così come è stato licenziato dalla Conferenza dei Capigruppo, vi saranno numerosi interventi e numerose richieste di modifica, cui seguiranno conseguentemente occuperà quindi per un tempo non brevissimo. Subito dopo l'esame e l'approvazione del calendario, come abbiamo appreso, è prevista la discussione del decreto-legge contenente le misure per fronteggiare la crisi finanziaria in area euro in relazione alla grave situazione greca.

sul calendario, contenente l'inclusione del provvedimento sulle intercettazioni telefoniche. La nostra è una richiesta di buon senso, che le viene rivolta nell'interesse del Paese e del Parlamento. Mi auguro che gli

si tratta di un provvedimento che tenta di mettere al riparo la sicurezza dell'economia internazionale, quindi ha una valenza sovranazionale,

Nulla osta dal nostro punto di vista, dopo aver accolto i suoi inviti nei giorni scorsi a differire la richiesta, a discutere prima il provvedimento che riguarda le vicende finanziarie ed il prestito alla Grecia, su cui c'è condivisione, e poi il calendario. Non abbiamo

Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte dell'area euro assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010. Come è noto, le linee di intervento messe in atto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea nelle riunioni del 2 e del 9 maggio mirano a fronteggiare la situazione di crisi finanziaria che si è manifestata negli ultimi mesi sui mercati internazionali, che ha colpito in modo specifico la Grecia e minacciato altri Paesi dell'area euro. Una crisi che il nostro Paese è chiamato in prima linea ad affrontare, costituendo una minaccia alla stabilità complessiva dell'eurozona.

dicevo, questa è una crisi che il nostro Paese è chiamato in prima linea ad affrontare, costituendo una minaccia alla stabilità complessiva dell'eurozona, uno spazio monetario ormai unificato che non conosce più confini nazionali e politici e che impone azioni coordinate e congiunte tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea. È in questo scenario che si è delineata la necessità di far fronte al grave squilibrio economico e finanziario, che ha riguardato in particolare la Grecia ma che investe anche altri Paesi europei. La 5a Commissione ha approvato il decreto all'unanimità, accogliendo del pari all'unanimità un emendamento del Governo che inserisce in norma la sostanziale ratifica dell'Accordo dell'8 maggio Nella riunione del 2 maggio scorso, il Consiglio europeo ha stabilito l'istituzione di un meccanismo di prestiti bilaterali per un ammontare di 110 miliardi di euro (di cui 30 a carico del Fondo monetario internazionale) per permettere alla Grecia di coprire il proprio fabbisogno finanziario. La concessione di questa linea di credito è però vincolata al rispetto di un programma che la Grecia, di concerto con la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale, si è impegnata ad attuare attraverso una manovra di aggiustamento degli interventi tesi a favorire la competitività e delle misure che regolino i mercati finanziari. Il decreto-legge in esame autorizza il Governo a realizzare le operazioni di sostegno finanziario a favore della Grecia concordate a livello internazionale. autorizza l'erogazione di prestiti sino al limite massimo complessivo di euro 14 miliardi e 800 milioni nel triennio. Ricordo che l'ammontare del contributo di ciascun Paese è determinato sulla base della quota di partecipazione al capitale della Banca centrale europea, per l'Italia pari al 18,42 per cento. L'articolo 2, comma 2, del decreto provvede ad autorizzare l'emissione di un ammontare di titoli a medio lungo termine espressamente in deroga al limite massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla legge finanziaria 2010. All'interno dell'eurozona si è maturata, dunque, la consapevolezza di dover promuovere un'azione condivisa a tutela di una stabilità finanziaria d'insieme, che sottende la comune volontà di contribuire, attraverso prestiti bilaterali coordinati, all'attivazione di un programma a sostegno della Grecia. Ritengo, tuttavia, fondamentale evidenziare l'esigenza che il programma di sostegno alla Grecia non si consideri soltanto come una misura straordinaria di assistenza finanziaria ad uno Stato gravemente a rischio di fallimento. Deve invece considerarsi come un'opportunità politica per assumere più profondamente la consapevolezza di una responsabilità comune, per migliorare gli strumenti operativi a tutela della stabilità finanziaria europea. A tale proposito, vorrei ricordare anche che l'Italia ha sostenuto la creazione di un Fondo di stabilizzazione nell'ambito dell'Unione come strumento immediato di gestione delle situazioni di crisi dei Paesi membri, adottato dal Consiglio europeo il 9 maggio scorso, con l'obiettivo di preservare la stabilità, l'unità e l'integrità dell'eurozona. È evidente dunque che in questo momento storico l'Unione europea e l'Italia, in particolare, hanno colto l'occasione per rafforzare le linee di una politica economica comune, per realizzare, con un moto di orgoglio comunitario, una coesione economica, sociale e territoriale più concreta ed efficace, in grado di rafforzare l'Europa e la stabilità dell'euro sui mercati internazionali. Forte coordinamento delle politiche economiche, quindi, a sostegno della Grecia e non solo. La crisi ha avuto il merito di costringere i Governi dell'eurozona ad approfondire il coordinamento delle politiche di bilancio, a mettere in moto procedure di sorveglianza dei conti pubblici, a mettere in gioco strumenti che costituiranno un modello per fronteggiare altre emergenze future. Il percorso verso una politica di integrazione è oggi più che mai una priorità che richiede, da parte di tutti, coincidenza di intenti, collaborazione delle istituzioni nazionali e fermezza nelle decisioni dei Governi. in questa situazione di grave crisi, il Governo italiano ha dimostrato una coscienza seria e rigorosa che ha evitato al nostro Paese di naufragare sotto i colpi della tempesta economico-finanziaria che ha sconvolto il vecchio continente. In quest'ottica va letta anche la nuova manovra a cui il Governo, in questi giorni, sta lavorando e che sarà oggetto dell'odierna riunione del Consiglio dei ministri. I tagli colpiranno a 360 gradi tutto il comparto pubblico. Il contenimento della spesa nazionale servirà ad assicurare anche la stabilità monetaria europea dell'eurozona, d'altronde in linea con le manovre che stanno attuando tutti gli altri Stati membri. Si tratta di una manovra di *austerity* e rigore che mira a ridurre i costi pubblici, ma che non trascura quella crescita necessaria al rilancio del *welfare*, dell'Italia e dell'Europa intera. In tal senso, l'approvazione di riforme incisive che producano effetti sostanziali e duraturi sulla dinamica della spesa corrente impone uno sforzo di elaborazione e di sintesi da parte del legislatore che sappia coniugare le esigenze del risanamento con l'obiettivo di salvaguardare comunque uno Stato sociale, efficiente e produttivo. La sfida che si prospetta è assai grande. È il tempo di avviare il Paese verso un percorso che assicuri la realizzazione concreta dei diritti sociali fondamentali, operando nella consapevolezza che il rigore nell'utilizzo delle risorse collettive e l'equità nella distribuzione del carico fiscale, modulati verso un'imprescindibile prospettiva di crescita, consentiranno al Paese di consolidare la propria posizione negli scenari competitivi internazionali. Come forze parlamentari, nel percorso che ci attende, di cui il presente decreto è solo il primo passo, abbiamo il dovere inoltre di rispondere all'appello opportuno del Capo dello Stato che ci invita ad un rigore e a un senso di responsabilità al di sopra degli schieramenti di parte. Ci troviamo di fronte ad uno sforzo impegnativo nel presente per un risultato significativo nel futuro.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, se c'è un termometro che indica l'importanza dell'Unione europea e della moneta unica sono le imprese italiane che - di fronte all'altalena dell'euro - non riescono ad adeguare i loro piani produttivi e faticano a mantenere i livelli di vendita con ripercussioni pesanti sia sullo sviluppo che sul mantenimento dei livelli occupazionali. Non sembrano affatto toccati dai problemi dell'economia reale, invece, gli speculatori, alcune banche e istituzioni finanziarie che, lasciate senza regole dalla politica, hanno generato e continuano ad ingenerare una caduta economica che imprese, lavoratori e intere Nazioni, come la Grecia, si trovano a dover pagare. Questi grandi operatori finanziari, come li chiama qualche giornalista, hanno spacciato, e si sono perfino fatti certificare, titoli senza valore senza valore come se fossero i migliori investimenti del mondo. Non lo erano e, alla fine, a pagare il conto salatissimo è stato chi lavora per produrre ricchezza vera. Ha detto bene il ministro Tremonti nell'informativa alla Camera dei deputati del 6 maggio scorso sulla situazione della Grecia: «Non è questa una seconda crisi che è arrivata. È solo la stessa crisi che è continuata e si è trasformata, passando dai debiti privati ai debiti pubblici e, così, scalandosi su scala globale». La soluzione a questo problema l'ha individuata ancora il nostro Ministro dell'economia: «Rimossi i confini economici, non si possono più far valere ora i confini politici». La soluzione, cioè, va ricercata in una maggiore coesione politica, in nuove, severe regole condivise da tutti gli Stati europei, sull'esempio di quelle varate negli USA venerdì scorso dal presidente Obama. Insieme ad altri otto senatori della maggioranza avevo presentato, nell'aprile 2009, una mozione con la quale esortavo il Governo ad agire in sede europea perché venisse istituita una *bad* *bank* dove concentrare ed isolare i titoli tossici e perché fossero emanate regole per eliminare il gigantesco conflitto di interessi tra le agenzie di *rating* e le società di emissione dei titoli. Proponevo così di affidare al Fondo monetario internazionale la certificazione di tutti i titoli trattati a livello internazionale. Infine, ma non è meno importante, si chiedeva di considerare l'ipotesi dell'istituzione di un tribunale internazionale per i crimini economici. Purtroppo la mozione è rimasta sulla carta: è passato un anno e nessuno ha inteso considerarla in alcuna delle sue parti. Ed oggi ci troviamo in un crinale che ci obbliga a scrivere delle regole quel tribunale, prima o poi, la storia forse lo insedierà e il suo giudizio sarà duro. Altri Paesi, dall'Irlanda alla Spagna e al Portogallo, sembrano sul punto di dover chiedere alla Comunità europea quello che stiamo concedendo alla Grecia. Se ciò avvenisse, come potremo imporre ai cittadini e alle imprese nuovi sacrifici per colmare i buchi creati dai finanzieri se, ancora oggi, costoro si dividono, come fossero un guadagno delle proprie azioni, gli aiuti statali? È questo che io vado domandandomi. La quota dell'Italia del prestito, per quanto in un primo tempo, comporti un esborso di 5,5 miliardi di euro, è forte: 14 miliardi e 800 milioni complessivi in tre anni. La Grecia, per ottenere questi denari, si sta fortemente impegnando per rientrare nei parametri determinati dall'Unione, ma la situazione sociale del Paese è difficilissima. Lo vediamo tutti i giorni. I *media* ci rappresentano quotidianamente lo stato in cui vive quel popolo. È stato detto che forse la Grecia non ce la farà a stare dentro le condizioni onerose del credito. Io non penso che il prestito sia un cappio per Atene. Se così fosse, dovremmo ripensarlo, perché ciò che dobbiamo fare è gettare le basi per un nuovo sviluppo in tutta Europa, a partire proprio dall'evento Grecia. Salvare la Grecia vuol dire salvare l'Europa. È una scelta, non un destino ineludibile. Se noi scegliamo di salvare la Grecia dobbiamo, una volta per sempre, comprendere che tutti i Paesi europei debbono rinunciare alla tutela esclusiva dei propri interessi e guardare più lontano. Per uscire davvero dalla crisi, infatti, occorre che le imprese tornino a produrre ricchezza, che siano sostenuti i consumi dei cittadini, che i bilanci degli Stati non siano più ostaggio delle banche che ne finanziano gran parte del debito. Questo, però, va accompagnato da regole che fissino i ruoli dei diversi soggetti economici perché ciascuno torni a svolgere il proprio ruolo in maniera più coerente e veramente solidale e - sottolineo il termine - insieme con gli altri. Se tutto questo nostro dibattito si risolvesse semplicemente con l'approvazione di un prestito, per quanto questo cada in un momento non facile per la nostra economia e costasse qualche sacrificio, non sarebbe davvero un grande problema. credo che dobbiamo cogliere questa occasione per prefigurare un progetto per l'Europa che al momento non si vede. L'Europa ha bisogno una nuova *leadership* politica che permetta la ripresa economica, sociale, finanziaria ed etica dell'Unione, e non di un organismo che in mille piccole decisioni quotidiane fa pesare gli interessi degli Stati più forti. Non è questa l'Europa unita a cui avevano pensato De Gasperi, Adenauer e Schuman. Questa è l'Europa che non c'è. Non c'é ancora. Perché se non ci possiamo permettere il fallimento della Grecia, non è nemmeno pensabile il fallimento del progetto politico europeo che riporterebbe i Paesi membri in una situazione di balcanizzazione economica e monetaria nonché di forte soggezione di fronte ai grandi soggetti emergenti nella scena mondiale, a cominciare dalla Cina e dall'India. Il progetto dell'Unione deve continuare a consolidarsi e la politica di integrazione dei nuovi Paesi non può prescindere dall'irrobustirsi della *governance* politica. Il senso del voto favorevole che qui esprimo rispetto alla decisione di sostegno della Grecia assunta il 25 marzo dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione è che l'Europa non sia considerata solo la zona euro, ma il soggetto capace di progetti e regole nuove per uno sviluppo solidale di un continente che può essere ancora un esempio di democrazia e un faro di libertà. Vi ringrazio per l'attenzione.

Debbo manifestare la mia e la nostra soddisfazione per la decisione del Governo e, in particolare del Presidente del Senato, di consentire che la votazione, che immagino unanime, su questo decreto possa precedere la fase dello scontro che inesorabilmente ci sarà sul calendario dei lavori in rapporto all'esame del provvedimento sulle intercettazioni. Questo decreto è necessario per tradurre in atto gli impegni che abbiamo preso

forse nei confronti della Grecia come sistema europeo siamo stati troppo generosi, abbiamo chiuso troppi occhi nel passato e forse, avendo accumulato un grande ritardo nel mettere in atto un provvedimento di emergenza, oggi possiamo dire, in rapporto ai contenuti del provvedimento di emergenza, che forse compensa la cecità di un tempo e gli sconti esagerati che abbiamo fatto con un carattere oneroso del provvedimento stesso al nostro esame rispetto alla Grecia che avrebbe potuto, forse, essere mitigato. Tuttavia, signora Presidente, vogliamo cogliere tale occasione per avviare anche in questa sede, nel Parlamento italiano - la sede più giusta - il dibattito sulle misure necessarie per uscire da una crisi drammatica come quella nella quale noi, assieme al resto dell'Europa, siamo precipitati. Qual è, colleghi, la posta in gioco? Non credo sia esagerato dire che si sta decidendo e si deciderà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sulla riscrittura della Costituzione materiale europea. Non facciamoci fuorviare dalle polemiche sulla speculazione internazionale. È verissimo che essa è all'opera ed è ovvio che va contrastata con tutti i mezzi nel tentativo, come si dice, di fargliela pagare - se ci riusciamo - agli speculatori, ma se ci si concentra solo sulla speculazione si seminano illusioni e si commettono degli errori. Illusioni, come quella che ha portato a dire, nei giorni immediatamente successivi l'accordo europeo, che con quel piano di interventi straordinari di garanzia di garanzia eravamo fuori dalla crisi. Non è assolutamente vero, perché la crisi ha a che fare con grandi contraddizioni macroeconomiche che restano del tutto irrisolte e non possono, per definizione, essere risolte da interventi straordinari. Errori, come la decisione unilaterale tedesca di vietare le vendita allo scoperto, a proposito della quale vorrei solo ricordare, a titolo di

Lo ricordo perché nei giorni scorsi è stata ventilata su tutti i giornali l'ipotesi che questo decreto venisse usato - e non lo è stato: ne voglio dare atto al Governo - per veicolare un emendamento che

in ogni caso, non ne sentiremo parlare più. In conclusione, se la posta in gioco è la futura Europa (di questo stiamo parlando), ciò di cui c'è bisogno sono niente di meno che due cose. anzitutto una scelta di posizionamento dell'Italia nel confronto, che è in atto alla dimensione europea, tra le due possibili linee di definizione di una nuova Costituzione materiale europea

è quella di un nuovo salto del processo di unità politica dell'Europa, ma costruito attraverso la definizione delle sedi, degli strumenti e delle scelte di politica economica e di bilancio alla dimensione europea. È la strada che preferiamo, perché è quella che consente di aggredire, a partire da una gestione europea del debito pubblico europeo,

ha consistenti possibilità di essere intrapresa), volta invece ad adottare una soluzione che, certo, fa fare un salto nel processo di unità politica dell'Europa, ma che lo realizza attraverso vincoli costituzionali, per esempio quelli sul deficit adottati recentemente dalla Germania nella sua Costituzione. La prima scelta da fare è questa: dove è il confronto in Parlamento per un atto di indirizzo nei confronti del Governo sul posizionamento da assumere in questo confronto europeo? Certo, stiamo discutendo del decreto Europa, ma l'occasione è straordinaria

La seconda cosa di cui la dimensione nazionale ha bisogno è niente di meno che un piano triennale per il rilancio della competitività del sistema Paese, perché solo un piano fatto di riforme strutturali è in grado di affrontare le ragioni per le quali l'Italia è così esposta alla crisi che stiamo vivendo. Questa crisi non nasce infatti dall'iniziativa degli speculatori, ma dal fatto che questi ultimi vedono che ci sono Paesi nell'ambito dell'area euro che non sono in grado prevedibilmente di onorare i loro impegni e, quindi, fanno il loro mestiere: speculano su questa scommessa. La situazione della Grecia è insostenibile da molto da molto tempo. Avevo raccolto dei dati per dimostrare tale affermazione, ma in pochi minuti non si può insistere su questo argomento e quindi li do per conosciuti. Su questo punto, in conclusione, a me sembra che, certo, ci vogliono atti come questo decreto; certo, ci vuole l'accordo europeo per mettere in campo i 750 miliardi di euro di cui stiamo parlando: queste queste iniziative sono assolutamente indispensabili, ma servono per prendere tempo. Il tempo per fare che cosa? Questa è la domanda cruciale. iniziative di riforma strutturale che vadano alla radice dei problemi delle grandi contraddizioni macroeconomiche alla base di questa crisi e il tempo necessario per accompagnare queste riforme di struttura alle iniziative immediatamente efficaci che sono necessarie per ridurre la spesa pubblica e, se possibile, per trovare nuove fonti di entrata. Questi interventi immediati, straordinari, di urgenza per ridurre la spesa pubblica e, quindi, per svolgere un'azione di riequilibrio nei conti pubblici italiani hanno però un senso e appaiono efficaci in quanto si collochino dentro quel disegno di mutamento strutturale di cui ho parlato prima. C'è un punto sul quale noi dobbiamo prendere una determinazione conclusiva; il Governo si deve porre e deve fornire una risposta efficace alla seguente

Se il Governo sostiene ancora questa tesi - le misure di emergenza, per carità, le possiamo vedere e discutere, molte di quelle le possiamo anche condividere - dobbiamo avere la consapevolezza che non stiamo affrontando la crisi, non stiamo ricollocando il sistema Paese dentro dentro una prospettiva di rilancio delle sue capacità competitive. Altra cosa è discutere di ognuna di queste misure immediate, straordinarie e di emergenza nel contesto di cui ho detto. Nei giorni scorsi e nel dibattito in Commissione ho avuto modo di ricordare che, ad esempio, ci sono tre interventi di tipo strutturale che a me paiono assolutamente essenziali: uno sul versante della applicazione della legge Brunetta-Ichino (una delle poche leggi di riforma che abbiamo adottato con un voto largamente condiviso) per fare in modo che le misure di rinvio di spesa, di rinvio dei rinnovi contrattuali o le misure di cui si sta parlando, come il blocco del *turnover*, siano inserite all'interno di questo grande disegno di radicale rivoluzione nell'assetto della pubblica amministrazione italiana. italiana. Si può essere d'accordo o meno sulle misure di blocco, di emergenza, ma esse si collocano dentro un disegno comprensibile e, a mio avviso, il Paese - ed in esso il Partito Democratico - dovrebbe essere disponibile ad un confronto di merito che conduca ad un esito favorevole. riguarda il fisco, certamente bisogna intervenire anche con misure di emergenza, perché bisogna trovare le risorse necessarie per far fronte ai rischi di collasso, ma dovremmo dovremmo adottare una politica fiscale finalmente generosa nei confronti delle risorse fondamentali presenti nel Paese, che sono le potenzialità per lo sviluppo: ad esempio una differenziazione drastica delle aliquote di prelievo sui redditi da lavoro delle donne rispetto ai redditi equivalenti dei lavoratori maschi. Sono convinto che questa misura darebbe un respiro alle misure di emergenza sul fisco, ne trasformerebbe in modo consistente la qualità e darebbe il segno che stiamo finalmente lavorando al cambiamento del Paese. La terza misura sono le liberalizzazioni:

che, nel giro di dieci anni, con accorte, radicali e coraggiose liberalizzazioni, in particolare nel settore dell'energia, in quello delle libere professioni e delle prestazioni di servizio di tipo intellettuale, potremmo recuperare 14 punti di competitività. La maggioranza porta in Aula un disegno di legge di riforma della professione forense che farà perdere ulteriori capacità di competitività al sistema delle libere professioni in Italia rispetto alle prestazioni fornite da altri Paesi, tant'è che la bilancia commerciale in questo campo del nostro Paese

nel funzionamento del sistema economico italiano? Vogliamo procedere alla separazione proprietaria di Snam Rete Gas dall'ENI? C'è un decreto che aspetta di essere attuato, i Governi di centrosinistra si susseguono a quelli di centrodestra,

vostra pazienza. Volevo solo dare il segno che per noi il voto favorevole su questo decreto avrebbe dovuto e potuto, e potrebbe ancora essere, il primo atto positivo,

perché, se non ci fosse, saremmo in condizioni un po' più difficili, e meno male che qualcuno accettò e facilitò l'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio. quindi, la soluzione al dramma e al pericolo cinese è stata tutta una politica introvertita e localista: «Dio, Patria e famiglia», dice espressamente il Ministro dell'economia. Credo però che oggi ci rendiamo conto che, in realtà, o riusciamo a reggere con l'esportazione e l'internazionalizzazione, oppure, in attesa che aumentino i consumi interni, possiamo anche chiudere bottega! modo, ci è stato detto per due anni che la crisi era psicologica e che quindi bastava un po' di fiducia, bastava aumentare i consumi per risolvere il problema, e così siamo andati avanti con i soliti

Si è continuato poi, com'è già stato ricordato, con il totem assoluto secondo cui in tempo di crisi non si fanno riforme. Si è continuato anche a non vedere come la questione demografica, demografica, nel nostro Paese come in molti altri, sia ormai rilevante in termini di perdita di competitività; eppure non c'è stato verso neanche di legalizzare la massa di lavoratori immigrati che tutti sappiamo che ci sono

È arrivato ora il momento della verità. Affronterò oggi tre o quattro questioni europee, rinviando poi al dibattito sulla manovra qualche verità italiana.

Vogliamo dire che la Grecia ha mentito sulle cifre e sui conti che ha trasferito a Bruxelles, mandando delle cifre letteralmente taroccate?

propose un Regolamento per affidare ad Eurostat un potere di *audit* sulle statistiche nazionali, quel Regolamento fu respinto da tutti gli Stati europei, perché nessuno voleva sottoporre le proprie cifre a controllo?

che non è una questione di speculatori (peraltro il mercato fa il suo mestiere), ma è una questione di scelta politica dei Governi, di quelli che ancora pensano all'Europa delle Patrie invece che alla Patria europea, illusi che l'autonomia nazionale, il fatto che nessuno metta il naso, in questo caso, nei nostri conti, sia un toccasana chissà verso dove. In realtà, ci ha mandato contro un muro ed è l'ennesimo costo della non Europa. Europa. Al di là di questo provvedimento tampone tardivo, al di là dell'intervento straordinario di 750 miliardi deciso il 9 maggio con grande euforia, le Borse e i mercati sono rimasti euforici per 24 ore, credono: non ci credono perché se, accanto a questa ingente massa di denaro, non c'è anche un rafforzamento istituzionale dell'Europa politica è chiaro che la fiducia non può essere recuperata.

fin quando in una notte sola il nostro Ministro fortunatamente è diventato eurofilo; ma il problema adesso è andare avanti su questa strada. Non vi sembri una pura provocazione, ma non è proprio pensabile una moneta unica basata su un bilancio dell'1 per cento del prodotto interno lordo. Il bilancio europeo è di 110 miliardi e abbiamo adesso fatto un fondo straordinario di 750 miliardi. È chiaro che tutto questo, senza un rafforzamento istituzionale, non dà fiducia a nessuno; non dà fiducia a nessuno non solo la mancata prospettiva di una crescita nei vari Paesi, ma il fatto che la costruzione, così come prevista, funziona in acque normali, in tempi normali, non è attrezzata in tempi di tempesta. Per dirla fuori dai denti, o arriviamo al Ministro del tesoro europeo, con relativo aumento del bilancio (può essere una federazione *light*, può essere una federazione che lascia fuori alcuni grandi settori dove i nostri sistemi sono diversi: penso al *welfare*, piuttosto che alle pensioni), o non è proprio possibile pensare che un'entità con questo bilancio dia sufficiente fiducia ai mercati, che infatti non ce l'hanno avuta (anche oggi le borse mi pare siano al profondo rosso). signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, credo che la strada vera non sia più quella funzionalista: oggi, o c'è il coraggio del rilancio del progetto europeo in termini politici (perché è la politica che salverà l'economia e la moneta e non l'inverso) verso quello che noi radicali amiamo chiamare, con Spinelli e persino con Winston Churchill (pensate un po'), gli Stati Uniti d'Europa quello che noi chiediamo è l'Europa delle Patrie - oppure tutto il resto sarà caro, carissimo, penoso per i cittadini, ma non ci farà riuscire a riconquistare un posto posto nello scenario globale, nello scenario internazionale, che pure va mutando sotto i nostri occhi con una velocità straordinaria. signor Vice Ministro, mi piacerebbe che, come in tempi passati, il nostro Paese fosse la bandiera, la punta di lancia per una ripresa e una rivitalizzazione del progetto federalista europeo. Non abbiamo scelta, credo che gli episodi di questi giorni e di queste settimane ce lo dimostrino in modo evidente. Certo, siamo circondati da altri Paesi meno disposti, ma penso che una convinzione ed una forte determinazione anche del nostro Paese potrebbero invece e finalmente cambiare il corso, che è un corso di declino delle varie Patrie europee, un corso di declino di quello che è stato il sogno non solo dei padri fondatori e delle madri fondatrici, ma di tutti coloro che hanno a cuore la promozione di entità geografiche non solo basate sull'economia, ma anche sulla promozione di legalità, democrazia e Stato di diritto.

i greci ricordano bene la frase di due sole parole pronunciata da Harílaos Trikoupis al Parlamento ateniese il 10 dicembre 1893:

Senza mezzi termini, l'allora Primo ministro comunicò l'insolvenza dello Stato nei confronti dei creditori esteri. Un precedente così remoto non significa quasi nulla, anzi l'Italia non è mai stata insolvente, a differenza della Germania come diretta conseguenza della riforma monetaria del 20 giugno 1948. Ma non per questo lo Stato tedesco, che sta maturando la convinzione di uscire dall'euro per ritornare al marco, è ritenuto meno affidabile di quello italiano. Condivido molto poco di quello che è stato detto dai senatori prima di me, ossia gli speculatori fanno il loro mestiere: sono i Governi che non fanno il proprio mestiere. Voglio ricordare che la crisi è datata luglio-agosto 2007, quando scoppiò lo scandalo dei *subprime*, delle agenzie di *rating* e della creazione del danaro dal nulla; la responsabilità dei banchieri, delle banche centrali colluse con le agenzie di *rating*. Voglio ricordare che, all'interno delle agenzie di *rating*, ci sono le stesse banche le quali, quindi, si fanno emettere pagelle per speculare su determinati titoli e su determinate valute. Qualche giorno fa il presidente della BCE, Trichet, ha detto che è necessario procedere con cautela nell'imposizione di un eventuale tasso sulle banche e ha ribadito che le divergenze nelle regole contabili a livello globale sono motivo di preoccupazione. Qui le banche, che hanno prodotto la crisi, sono preoccupate: i governatori centrali delle banche centrali, che non hanno fatto nulla per evitarla, sono preoccupati e coloro che subiscono gli effetti di una crisi sistemica senza precedenti che cosa devono dire? Mi auguro che non ci sia quella grande ribellione che scoppiò nella Francia del 1789, perché davvero la misura è colma. Noi diamo 750 miliardi di euro agli speculatori: noi armiamo i fucili, dandoli a basso costo, per fucilare l'euro. È quello che sta avvenendo. Da quando ho messo piede in questo Senato continuo a ricordare la responsabilità di quelli che sono distratti. Ho parlato anche di due tipi di corruzione, una economica e un' altra ideologica, che è quella più grave. Voglio ricordare che, dall'inizio della legislatura, abbiamo denunciato speculatori, affaristi e faccendieri che vanno a braccetto con gli Esecutivi, foraggiandoli direttamente o indirettamente, sia con ingenti risorse economiche che con i loro dirigenti più influenti. Andiamo a vedere da dove viene Timothy Geithner, il Segretario al tesoro americano, buono per tutte le stagioni. Andiamo a vedere Goldman Sachs, quella banca d'affari che ha erogato 3 miliardi di euro per finanziare tutti, ossia istituzioni, giornali e giornalisti. Voglio ricordare anche Ezra Pound a questi gnomi dell'alta finanza, che pretendono che i governi democratici svolgano la funzione di maggiordomo dei loro esclusivi interessi, dei loro *desiderata*. Ora che la crisi è sotto gli occhi di tutti, signori della maggioranza, signor rappresentante del Governo, dopo che l'avete occultata per ventiquattro mesi additando come anti-italiani tutti coloro che non vedevano l'ottimismo di facciata, ma una falcidia di posti di lavoro, una distruzione di ricchezza, una grave recessione: ora quindi che vi accingete ad una manovra lacrime e sangue a carico delle famiglie, occorre prendere decisioni imposte dalla gravità della situazione economica. Voglio citare il presidente degli Stati Uniti, Obama, che è riuscito a far approvare, nell'ostilità dei grandi magnati che governano i destini del mondo,

che pure ha gravissime responsabilità per avere ritardato gli aiuti alla Grecia, hanno adottato provvedimenti doverosi, perché la speculazione non la si deve finanziare. Non si può permettere che vengano utilizzate utilizzate le vendite allo scoperto per fucilare i Governi democratici e la sovranità degli Stati: non lo possiamo permettere.

i più fedeli esecutori dei banchieri alla Cassa depositi e prestiti, che gestisce 200 miliardi di euro di sudatissimi risparmi. Il Presidente degli Stati Uniti ha proposto una nuova tassa sulle responsabilità della crisi economica da imporre alle maggiori società finanziarie americane salvate dalla recessione con il denaro pubblico. Anche Dominique Strauss-Kahn ha accolto con grande favore l'annuncio, mentre gli istituti bancari si preparano a dare battaglia, come in Italia - tante sofferenze - e si accingono a mettere nuove commissioni a carico degli utenti e dei clienti, a lesinare il credito e a fare una gestione del credito del risparmio con criteri clientelari. L'ho detto altre volte a chi vanno dati 3 o 4 miliardi: non a chi li vuole utilizzare per attività produttive, ma agli amici degli amici, come nel caso I contorni della crisi sono analoghi a quelli già visti nel dopo Lehman: una forte contrazione della liquidità sui mercati finanziari: una contrazione degli scambi sui titoli di Stato: fuga dalle azioni, che continuano ad essere il mercato più liquido; maggior margine di garanzia dei clienti; liquidazione delle posizioni da parte degli *hedge fund*, ossia quegli investitori più rapidi a percepire i cambiamenti degli scenari; ricorsi frequenti di prestiti alla BCE (all'1 per tassi interbancari, come pure Euribor e Libor, in aumento, a dimostrazione che tra le banche cresce la diffidenza a prestarsi denaro vicendevolmente;

514 punti con la Grecia. E mentre il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, che ha portato a processo alcune banche per la vendita delle scommesse, i derivati, al Comune di Milano - voglio ricordare che anche Roma non è immune, anche se nessuno ne parla (3,6 miliardi di euro) - ha messo in guardia sui rischi della bomba derivati sugli enti locali, pari ad oltre a 35 miliardi - ciò è emerso anche nell'indagine conoscitiva che abbiamo fatto come Commissione finanze - la distratta Banca d'Italia comincia a pubblicare i dati sui CDS, i *credit default swap*, in pancia agli istituti di credito italiani, così virtuosi da avere qualcosa come 376,2 miliardi di dollari comprati e 387,1 miliardi di I giochetti e le scommesse dei banchieri italiani, analoghi a quelli effettuati dagli altri banchieri biscazzieri che acquistano questi CDS, contratti con cui si assicura il rischio di fallimento di un emittente di titoli, contribuiscono a portare alla rovina l'economia reale, a picco la stabilità dell'euro e della cosiddetta *old economy*. Il Governo per la manovra di lacrime sangue che sta preparando, invece di tassare i soliti lavoratori e pensionati - alla fine pagheranno sempre gli stessi - potrebbe trovare buona parte della copertura adottando

risparmio il differenziale delle virtuose banche italiane, che praticano i mutui ad uno 0,59 per cento in più rispetto alla media europea. europea. Le banche italiane sono stabili, ma quella stabilità gliel'abbiamo pagata noi, i correntisti e le piccole medie imprese, a rate, da decenni, con il consenso distratto della politica.

Ma ci rendiamo conto o no che queste agenzie emettono giudizi in conflitto di interesse,

che ha definito il rapporto di Moody's "assolutamente infondato". Infondato perfino per la terza sorella del *rating*, che è Fitch. Fitch. Su queste questioni non bisogna più scherzare, perché noi siamo seduti su una polveriera: per tre anni non ce ne siamo accorti

cioè la tassa sulle speculazioni. Anche questa è una misura che si può prendere e almeno se ne dovrebbe far carico il Governo nell'ambito del G20. la tassa sulle banche. I banchieri hanno prodotto la crisi e sono loro che si aumentano i *bonus* e le prebende. Vogliamo ricordare il signor Profumo,

terminare desidero solo dire che, poiché il Governo ha fatto la politica dello struzzo e ha dissimulato una crisi che era sotto gli occhi di tutti, noi, probabilmente

nel triennio. Rivendichiamo il diritto di andare soli: meglio soli che male accompagnati.

stabilisce la partecipazione dell'Italia all'impegno europeo di erogare prestiti bilaterali alla Grecia per garantire stabilità finanziaria nella zona euro nel suo complesso. Quali sono i criteri di massima? Il primo è quello in base al quale le risorse necessarie al rispetto del programma verranno reperite attraverso emissioni di titoli di stato a medio e lungo termine. Per onorare nei tempi previsti il programma di sostegno finanziario alla Grecia, il Governo ricorrerà ad anticipazioni di tesoreria. Gli importi delle emissioni non saranno calcolati nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria: il limite verrà ridefinito dal Ministero dell'economia con le occorrenti variazioni di bilancio. I rimborsi del prestito confluiranno nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e gli interessi destinati al pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato. Fin qui, i criteri di massima. In fondo, però, di che cosa si parla? Si parla di deficit: di deficit della Grecia, di deficit di tutta l'area del Mediterraneo. Ciò comporta due ordini di ragionamenti: uno è spostato sul campo europeo (come è stato fatto anche negli interventi che mi hanno preceduto). mi hanno preceduto). Che cosa si intende fare a livello europeo, che idea si ha dell'Europa, dell'economia, della finanza e della *governance* economico‑finanziaria e fiscale ragionamento è nazionale ed è inquadrato nella manovra che oggi è in esame. L'eurosoluzione adottata per salvaguardare l'economia del vecchio continente da nuovi *crack* finanziari lascia però aperti ampi spazi di riflessione su cosa aspetta l'Europa nei prossimi anni. Si è affrontata un'emergenza - l'ennesima - e si è cercato di prevenire le aperture di nuove voragini. Si è però detto poco sulle politiche e sulle strategie di sviluppo e di rilancio dell'economia dei 27 Paesi che oggi aderiscono all'Unione europea e sul futuro di quel quasi mezzo miliardo di esseri umani che, se unito, è certamente in grado di affrontare l'estremo Oriente superpopolato e superproduttivo. Va detto che lo sconvolgimento che sta attraversando le economie europee non sarà così grave come il *crack* finanziario che si è aperto due anni fa, perché, fortunatamente, ogni Paese europeo sta mettendo in campo politiche di aggiustamento per evitare qualcosa di più grave, come può essere il crollo dell'euro. Non basta, però, perché se i deficit rimangono così alti, se la crescita e la competitività non ricompaiono, se le riforme strutturali non vengono implementate, se non si stringe sul fisco, allora il tunnel potrebbe il tunnel potrebbe essere molto lungo. Senza queste misure persisterà il rischio che la Grecia, ed eventualmente altri Stati, possano essere costretti ad uscire dall'Unione europea. Per quanto riguarda il nostro Paese, esso non è certo tra i peggiori d'Europa, ma i problemi ci sono e sono tanti. Serve un ampio ventaglio di riforme fiscali e una razionalizzazione del settore pubblico e del sistema delle tasse e della spesa, da conciliare con una politica d'investimenti

e, con la lucidità dimostrata dal ministro Tremonti, affrontare la realtà della nostra situazione economica. La nostra stabilità finanziaria oggi, come avviene in altri Paesi, è ancora fortemente minacciata dalla Grecia, ma è legittimo chiedersi se, superata l'emergenza ellenica, il nostro Paese possa fronteggiare la situazione

pensare soltanto alla voragine del debito pubblico, perché ciò equivarrebbe a perpetuare lo *status quo*: è universalmente riconosciuto, ormai, che senza la crescita il deficit non si combatte. Più concorrenza, meno burocrazia, alleggerimento del carico fiscale e, quindi, infrastrutture ed energia meno cara sono alcune delle priorità del nostro Paese. Il Governo ha dato ampie rassicurazioni in tal senso, mettendo in cantiere una riforma fiscale

dell'Unione. Il disegno di legge originale della moneta unica prevedeva che, prima o poi, questo salto sarebbe avvenuto e i mercati finanziari si stanno domandando se si tratta di un sogno oppure di una prospettiva realistica seppure non immediata. La crisi di fiducia che sta attanagliando l'Unione europea non può essere affrontata soltanto con meccanismi di intervento straordinario. Per la prima volta, dopo anni di sostanziale assenza dal dibattito, la Commissione dell'Unione europea ha risposto alla sfida, proponendo una riforma radicale del Patto di stabilità e crescita, riforma che dovrà poi essere affrontata dai Paesi per diventare operativa senza senza che, tuttavia, questo richieda una revisione del Trattato europeo. Quindi, lo scenario complessivo entro il quale muoversi è stato indicato con chiarezza dalla Commissione europea per rafforzare la *governance* nell'Unione europea. L'autentica novità è rappresentata dalla proposta di aumentare la sorveglianza sulle finanze pubbliche di tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione europea. Invece di inseguire gli avvenimenti, d'ora in avanti occorre anticiparli con una preventiva analisi di livelli

per la stabilità monetaria dell'intera area dell'euro. Saranno necessarie riforme incisive, tuttavia salvaguardando il modello di stato sociale che si è affermato in Europa nel secolo scorso e che, ormai, fa parte integrante della nostra civiltà democratica. Ciò significa assicurare a tutti i cittadini i diritti fondamentali, utilizzando le risorse collettive che si determinano con il riconoscimento unanime del valore oggettivo di una sana economia di mercato e, con una equilibrata distribuzione del carico fiscale, rendere nuovamente competitiva l'economia europea e quella italiana. Concludo con una frase ricordata dal ministro Tremonti nel suo intervento del 6 maggio scorso alla Camera dei deputati. Svolgendo la sua informativa il Ministro, richiamando l'etimologia della parola crisi, ribadito che in greco essa vuol dire discontinuità. Questa discontinuità può risultare positiva e costruttiva per l'Europa; però i Governi europei devono riconoscere l'urgenza di affermare maggiore coesione e di unità di intenti. a parlare il senatore Mascitelli, Signor Presidente, la farsa sembra finita. Il falso *slogan* berlusconiano secondo cui la crisi sarebbe da tempo alle nostre spalle non incanta e non inganna più nessuno. La crisi, signor Vice Ministro, è ancora tutta davanti a noi e minaccia addirittura il cuore dell'Europa, i fondi sovrani dei suoi Stati membri e la moneta comune. Il 6 maggio, pochi giorni fa, nella sua informativa sulla crisi economico-finanziaria in atto in Grecia e sulle possibilità di ripercussioni sulla stabilità dell'Europa, il ministro Tremonti dichiarava: «È ancora incognito quanto può accadere - stiamo parlando del 6 maggio - e sta accadendo nella fascia che va dal Baltico ai Paesi meridionali dell'Est Europa». Purtroppo non c'era nulla di misterioso nell'aggravarsi della crisi o, meglio, c'è, ma il problema riguarda più la politica che l'economia. Sulla Grecia si doveva intervenire da tempo. Già a partire dal 2005 la Commissione europea ed EUROSTAT esprimevano riserve circa la veridicità dei dati riportati sull'indebitamento e nuovi dubbi sulla copertura in relazione ai fondi fuori bilancio venivano presentati nel 2008. Si è, invece, tergiversato alla ricerca di un compromesso che salvasse capre e cavoli, che consentisse, da un lato, al Governo greco di preparare i tempi e le modalità degli inevitabili sacrifici e, dall'altro, alle banche di poter mettere in sicurezza i propri beni senza al contempo spaventare troppo l'elettorato tedesco e anche quello italiano nelle imminenti competizioni elettorali. Sappiamo tutti che il percorso di rientro del deficit della Grecia dal 14 per cento, con una continua discesa dal 2002, è quantomeno ambizioso: solo per questo anno la correzione del rapporto deficit e PIL dovrebbe essere di circa 5 punti dall'attuale 14 per cento. Il rapporto dovrebbe scendere sotto il 3 per cento nel 2014, cosicché le misure adottate rischiano di essere quantomeno poco realistiche.

Dopo anni di inerzia e anarchia finanziaria bisogna rendersi conto che l'euro rappresenta sì una garanzia importante, ma non è più da sola sufficiente. Occorre intensificare i controlli sulle finanze interne dei singoli Stati, rafforzare il coordinamento tra le varie economie dell'euro, introdurre politiche e procedure, liberalizzazioni e strumenti di *welfare* comuni. Signor Vice Ministro, abbandonare l'ipocrisia del falso europeismo. La Grecia ha un debito verso l'Europa di 236 miliardi di dollari, il Portogallo di 286 miliardi, l'Irlanda di 867, la Spagna di 1.100, l'Italia di 1.400; la Grecia deve 9,6 miliardi di dollari al Portogallo, che ne deve 58 alla Spagna, che ne deve 14 all'Irlanda. È un gioco di scatole cinesi del debito in cui alla fine tutti possono rimanere con in mano un cerino accesso. La Francia ha un credito verso l'Italia, che ha il più importante debito europeo, pari al 20 per cento del suo PIL.

non sta tanto nei prestiti che i 15 Paesi dell'area euro sono disponibili a concedere, che sono a tutti gli effetti prestiti bilaterali che andranno così ad aumentare ideficit pubblici anche dei Paesi più indebitati. Il problema non sta nel fatto che i prestiti concessi dai partner europei potrebbero rivelarsi anche un buon affare, come si dice nella relazione, visto che per loro il costo del finanziamento è di 2-3 punti percentuali inferiore rispetto al 5 che viene fatto pagare alla Grecia. Il problema principale, squisitamente politico, è nel segnale di scarsa fiducia che queste stesse condizioni, contenute nel decreto, comportano ed implicano. Oggi i Paesi europei con debiti molto alti, ma non soggetti alla speculazione, riescono ad indebitarsi a tassi pari a circa la metà di quelli richiesti alla Grecia. Allora la politica economica, se fosse veramente una politica economica europea, non dovrebbe allinearsi al mercato, se il suo obiettivo è quello di contrastare le aspettative destabilizzanti. Altrimenti le pratiche speculative trovano alimento nel comportamento e nella perdita di credibilità stessa delle istituzioni. Una seconda considerazione merita il sistema bancario europeo. Oggi la Banca centrale europea, attraverso gli strumenti di politica monetaria, è di fatto uno dei maggiori finanziatori dell'economia ellenica. Se domani il Governo greco dovesse dichiarare il *default* dei propri titoli pubblici o addirittura l'uscita dall'euro, il bilancio della BCE sarebbe il primo a risentirne. Le principali banche europee - lo ha ricordato poc'anzi il collega Lannutti

Sul caso della Grecia il ministro Tremonti ha dichiarato, sempre nella sua nota informativa alla Camera dei deputati, che sono emerse impressionanti e prima non rilevate asimmetrie informative. E a proposito di asimmetrie informative il Governo nel nostro Paese ha acquisito una sua particolare e peculiare esperienza. In Italia, infatti, si è passati dalla denigrazione delle statistiche ad una fase più subdola, quella di oscurare i numeri sull'andamento vero dell'economia che non piacciono al Governo. Ricordo che al convegno di Confindustria di Parma Berlusconi ha contestato le cifre fornite nella relazione introduttiva Governo. Ricordo che al convegno di Confindustria di Parma Berlusconi ha contestato le cifre fornite nella relazione introduttiva che documentavano - dati ISTAT alla mano il declino economico del nostro Paese, un calo cioè del 4,1 per cento del reddito *pro capite* degli italiani dal 2000 al 2009. Il Governo sostiene che l'Italia ha resistito meglio di altri all'impatto della crisi mondiale: per avvalorare questa tesi viene citato molto spesso il basso indebitamento delle famiglie e la forza del settore manufatturiero. Sul primo dato, non dobbiamo dimenticare che i risparmi in questione si sono assottigliati in questi due ultimi anni, come dimostra il calo dei consumi, e che le nostre imprese sono altamente indebitate e soffrono in misura sproporzionata della stretta del credito. Sul secondo dato, quello manufatturiero, i numeri riguardano principalmente le esportazioni manufatturiere del nostro Paese. A parte che è discutibile l'attenzione sulle sole industrie manufatturiere, quando ormai la parte preponderante dell'economia mondiale è costituita dai servizi ed il commercio mondiale in questo settore cresce quanto se non di più del manufatturiero, che, pur essendo importante l'esportazione, è sbagliato prendere la crescita dell'*export* come indice di competitività ignorando e forse volutamente ignorando - i dati sulle importazioni, che nello stesso periodo sono aumentate più delle esportazioni, peggiorando il saldo commerciale del nostro Paese. È un modo per taroccare i conti della nostra economia. Ma andiamo avanti. Giorni fa è arrivato dalla Corte dei conti il primo rapporto sul coordinamento di finanza pubblica. Due sono le novità. le novità. Il problema serio che si pone è soprattutto di prospettiva e riguarda la dinamica del PIL, che entro il 2012 si sarà ridotto in termini nominali di 130 miliardi di euro, il doppio della spesa per interessi sul debito; una caduta senza precedenti che rende certamente più difficile una programmazione di bilancio, soprattutto se tardiva. La seconda novità che ci comunica la Corte dei conti e che offre al Parlamento italiano una lettura diversa del ruolo giocato dai diversi livelli di governo nell'aggiustamento del bilancio dello Stato rivela che il contributo importante garantito dalle amministrazioni locali, il disavanzo di Regioni, Province e Comuni, è stato pari allo 0,4 per cento del PIL contro lo 0,6 previsto.

Ma poiché nella storia degli ultimi venti anni esso è stato attorno al 2 per cento, la differenza del 2 per cento equivale a 20-25 miliardi all'anno in più: miliardi all'anno in più: sarebbe stato necessario che il governo ci avesse detto già da tempo come immaginava di recuperare tali risorse nel nostro Paese, visto che i consumi intermedi - un altro dato che forse il Governo sottace - anche quest'anno sono aumentati di ben 6 miliardi di euro, anziché ridursi come il ministro Tremonti ci aveva promesso un anno fa. Nei prossimi giorni, signor Vice Ministro, avremo la possibilità di approfondire e giudicare le singole misure della manovra che il Governo sta predisponendo. Però una cosa è certa: i tagli della spesa non sono fatti sulla carta, sono reali. Si tagliano le persone, si tagliano in gran parte stipendi, o comunque soldi che alla gente non arriveranno più.

parlamentari - che la sforbiciata sugli enti inutili sia veramente coraggiosa e che i tagli ai costi della politica non siano solo uno specchietto per le allodole.

Dobbiamo abbassare le tasse perché non sono eque e ostacolano la crescita, ma non possiamo farlo se non passando attraverso riforme strutturali della spesa che il Governo non ha mai fatto e, forse, non è in grado di fare; lo dobbiamo fare attraverso l'eliminazione dell'evasione fiscale ma anche della corruzione e del clientelismo, che il Governo non ha mai condotto e che, forse, non ha intenzione di fare seriamente. Ma continuando a non fare nessuna di queste cose saremo obbligati a subire sempre più non tanto e non solo le speculazioni di cui anche oggi si sta parlando,

Vice Ministro, questa sta diventando una legislatura sì di grandi riforme, che noi della Lega spingiamo, ma anche una legislatura di grandi riflessioni ed interventi in campo finanziario ed economico

senza un controllo e una reale *governance* avrebbero probabilmente determinato degli scompensi e delle preoccupazioni per quanto riguarda la tenuta e la normalità della vita dei nostri cittadini, delle nostre famiglie e dei nostri lavoratori.

abbiamo visto le difficoltà di Paesi appena entrati nell'area euro come quelli baltici, che, di fronte a variazioni di incremento di PIL

recentemente in Grecia, ma che non hanno magari avuto quel riscontro sui *mass-media* e quella vetrina che invece ora c'è, forse perché la Grecia è più grande, forse perché questo fenomeno si sta ripetendo, forse perché purtroppo sono avvenuti fatti molto dolorosi con delle vittime assolutamente non responsabili e degli attacchi e delle strumentalizzazioni di lotte cittadine, non certamente democratiche che condanniamo totalmente. Dicevo che avevamo rappresentato queste preoccupazioni, questa necessità di *governance* economica

di un grande periodo di riforme strutturali, che chiediamo da tempo e che finalmente si sono avviate; mi riferisco al federalismo fiscale e al federalismo demaniale,

Grazie, sulle spese medie di funzionamento delle pubbliche amministrazioni - il periodo è quello dei primi anni del 2000, ma comunque in questi ultimi anni

che ha una spesa di funzionamento al netto degli interessi sul debito molto elevata, ed un indice di funzionamento standardizzato in base alle spese di funzionamento il più elevato possibile rispetto a tutti gli altri Paesi, sia a sistema federale - questo è certamente comprensibile - che anche a sistema unitario quali ancora noi siamo (ma presto ci sdoganeremo da questa classifica e da questo gruppo per passare a quello dei Paesi federali). C'erano quindi i presupposti strutturali ed organizzativi della struttura amministrativa e quindi di distribuzione della spesa del Paese, che in un sistema

dove c'è produzione di reddito e dove avviene il trasferimento delle risorse da parte dello Stato centrale. Interveniamo coscientemente e con convinzione su questo provvedimento,

riflettere sul fatto che, se non fossero accadute le cose che stanno accadendo in questi giorni e in queste ore, ci saremmo limitati ad apprezzare la decisione del Governo, magari registrando il fatto un po' anomalo che con questo provvedimento ogni Stato membro dovrà emettere titoli che si riverseranno su un sistema finanziario già debole, che riceverà quindi un sovraccarico di impegno e di lavoro.

le buone e positive decisioni assunte il 10 marzo e nonostante l'annuncio della costituzione di un fondo di ben 750 miliardi che doveva mettere al riparo l'euro e l'Europa dalla speculazione mondiale.

bilancio. Prendiamo atto dunque che l'euro non è in grado di difendersi da solo e questo è il punto di criticità più evidente a livello istituzionale e strutturale. Perché, però, accade tutto questo? Si dice che abbiamo fatto male ad allargare l'Unione a 27 Paesi, molti dei quali non rispettavano i parametri stabiliti il 31 gennaio del 1992 a Maastricht: può darsi. la BCE è debole, ancorché la sua creazione sia stata costituzionalizzata nella Carta di ogni Paese membro dell'Unione Europea: ma è debole perché non ha il potere di incidere sugli altri Paesi membri, ma soprattutto - e questo il mercato mondiale lo sa - perché non ha uno Stato sovrano dietro, con una sua finanza pubblica unica ed indivisibile. Tutto questo è vero

sistema. Per questo credo, signora Presidente, che siano maturi i tempi per ripensare l'euro: del resto, il senso del dibattito che prende avvio in questi giorni e che proseguirà quando il Governo presenterà la propria manovra finanziaria,

C'è il mercato. La speculazione è il mercato; quindi, è vano, è illusorio, è miope ed infantile prendersela con la speculazione nell'economia globalizzata: la speculazione sono le condizioni che detta di per sé il mercato. Ma se così è, se così è, siamo convinti della bontà e della tempestività del Governo che in queste ore sta discutendo e definendo una manovra per dare un segnale forte al mercato circa le intenzioni dell'Italia ed incoraggiamo

che ripensare l'euro in realtà significa ripensare alla costituzione materiale di Maastricht (lo diceva il senatore Morando, e io sono d'accordo con lui). Ma ripensare che cosa? Ripensare la religione di Maastricht, ciò che approvarono Grazie, penalizza, certamente il nostro è un Paese molto esposto sul debito pubblico; ma quest'ultimo non è il problema, è uno dei problemi. Se quel giorno a Maastricht, anziché quei cinque parametri, ne fossero stati individuati altri, probabilmente le condizioni del nostro Paese apparirebbero a tutti assai diverse e migliori rispetto ad una condizione vera del mio Paese che ancora oggi ha la consistenza in termini di risparmio più forte del mondo, il sistema bancario e finanziario più forte dell'Europa; un patrimonio pubblico in capo allo Stato italiano che non ha eguali in tutta Europa; la quantità di riserve valutarie che ci collocano oggi terzi al mondo dopo gli Stati Uniti e la Germania. Quindi, acquisendo il superamento dei parametri di Maastricht e andando verso il superamento della costituzione materiale dobbiamo avere questa avvertenza. Guardate che il fatto che fa i nostri BTP siano stati aggrediti al punto che in una sola giornata hanno perso il 2,5 per cento ci riporta al lontano 1992; ci riporta ad una condizione nella quale l'ambito storico era diverso (allora entravamo in una stagione terribile, Tangentopoli), ma come disse un Ministro allora scoprimmo che non poteva durare un Paese che produceva come l'Unione Sovietica e consumava come gli Stati Uniti d'America. Certo, non siamo tornati a sono però delle avvisaglie terribili, che ci devono mettere in condizione di reagire con grande forza, evitando di seguire l'esempio della Gran Bretagna, questo grande Paese che per me è una grande delusione, perché tirandosi fuori in questo momento

per salvare, attraverso sei nazionalizzazioni, sei banche che erano fallite, tirando fuori più di 400 miliardi di lire sterline), oggi sta dimostrando una evidente incoerenza. Noi dobbiamo percorrere con convinzione la strada lungo la quale i debiti e le debolezze non possano essere trasferiti dai singoli Stati all'intera Europa. Allora, il nostro contributo al dibattito in quale direzione occorre mirarlo? Dobbiamo chiedere con forza, da parte di tutti i Capi di Governo, di mettere mano finalmente ad una più incisiva politica di coordinamento delle politiche economiche dei 27 Paesi dell'Europa; dobbiamo immaginare una politica di coordinamento economico che metta al centro l'innovazione, la ricerca, le politiche del lavoro per aumentare la competitività del sistema italiano e di quello europeo, ponendo così le condizioni per fare ad un tempo un mercato unico, ma anche un'area di tasso di crescita significativo. Per questo anch'io credo che assieme ad una politica di rigore vada ripensata la necessità di avviare riforme strutturali, quelle riforme che vanno fatte ancorché oggi le condizioni finanziarie siano quelle che sono. Penso che il fondo di 750 miliardi sia una rete di protezione, ma credo che varrà di più la convergenza delle politiche economiche, per evitare così che una crisi contagi anche altri Paesi oltre quello greco. C'è la necessità, secondo la mia opinione, di riscrivere il Patto di stabilità e di crescita. Ciò che appare chiaro a tutti, collega Lannutti, è che dopo il fallimento del sistema finanziario americano, dopo aver registrato le responsabilità gravi delle banche d'affari americane, dopo aver resistito allo tsunami partito dagli Stati Uniti d'America, credo che dobbiamo che dobbiamo aver coscienza delle condizioni del mio Paese. Lo dico con simpatia al collega Lannutti, che nel 2005, in quanto rappresentante dell'associazione consumatori Adusbef e oggi come senatore continua a ripetere «i banchieri, i banchieri, i banchieri»: cerchiamo di porre un punto fermo, altrimenti ci prendiamo in giro anche tra di noi. Certamente i banchieri americani l'hanno fatta grossa (per dirla in termini volgari), perché hanno inquinato non solo quello americano, ma l'intero mercato finanziario internazionale. però in un Paese che oggi a consuntivo - possiamo dirlo - ha avuto la capacità di resistere senza che fossero necessari interventi statali, statali, ossia senza interventi di salvataggio da parte dello Stato nei confronti del proprio sistema bancario. Questa - collega Lannutti - è la storia vera del mio Paese, del nostro Paese. Non altro. Quindi, per piacere, non si confonda anche lei. Vada a leggere la storia di questo Paese, magari gli atti parlamentari del 1990, quando questo Parlamento approvò all'unanimità la legge di riforma del sistema che ha prodotto la condizione di oggi, ossia di avere in Europa il sistema bancario più resistente, più patrimonializzato e più forte. Altro che quelle fughe in avanti che lei compie, confondendo i banchieri americani, inglesi e italiani. Sono storie diverse - collega Lannutti - che non ci appartengono. Mi avvio alla conclusione, che cosa deriva l'ottimismo, o meglio il realismo del Governo Berlusconi. Noi siamo in una condizione migliore di quella che appare. Siamo un Paese che sta meglio rispetto a quello che appare. Certo,

se saremo in grado di praticare con coerenza e coraggio le giuste politiche, che sappiano coniugare il rigore al rilancio di una politica economica mirata a sciogliere gli annosi nodi strutturali che ci trasciniamo da molti anni, credo metteranno il mio, il nostro Paese, per i fattori di base a cui ho accennato poco fa, nelle condizioni di prendere il rimbalzo e di crescere più degli altri Paesi.

La mia replica sarà breve. D'altronde, l'intervento del senatore Grillo è stato quasi esaustivo sui temi che riguardano il dibattito in corso. Mi permetto sommessamente di osservare che non ho capito, e trovo contraddittoria, la posizione degli esponenti colleghi dell'Italia dei Valori, i quali sostanzialmente hanno affermato che questo provvedimento arriva troppo tardi e oggi, poi, che è arrivato votano contro. Ritengo che la logica saggia del "meglio tardi che mai" sia comunque sempre valida, anche in questa occasione. si tratta soltanto di un primo piccolissimo passo in un percorso e credo che in questo il dibattito ci abbia accomunato in molte parti. Anche le sue osservazioni, presidente Bonino, e quelle del senatore Morando hanno comunque ammesso che l'azione del Governo italiano in questo frangente è stata opportuna, positiva, puntuale e tempestiva. Condivido

della Costituzione materiale europea. Ce lo auguriamo tutti, perché tutti siamo convinti che serve una maggiore efficacia e una più penetrante politica europea. Siamo tutti convinti, presidente Bonino, che la speculazione è un effetto dell'attuale situazione ed è un errore farlo - considerata la causa di quanto sta succedendo sui mercati e nelle economie reali dei Paesi. Inoltre, siamo tutti convinti che per recuperare la fiducia dei mercati c'è bisogno di rafforzare la politica europea, di rafforzare l'azione dell'Unione europea e dei Paesi membri sulle politiche economico-sociali dell'intero territorio europeo. Io credo che l'Italia, come diceva poco fa il senatore Grillo, il nostro Paese, in questo contesto

meno grave riguardo al deficit, su cui altri Paesi hanno problemi più evidenti. Abbiamo un sistema produttivo ancora sano e solido, che i segnali di questo primo trimestre danno in faticosa ma comunque significativa ripresa. Abbiamo un sistema bancario che comunque, in questi due anni di crisi internazionale, ha tenuto ha tenuto senza ricorrere al contributo dello Stato. In questi due anni il Governo ha attuato, credo, politiche sagge. Certo, possiamo discutere su ciò che di più e di meglio si poteva fare, ma ritengo che il Governo abbia mantenuto la barra dritta sull'equilibrio dei conti pubblici e della finanza pubblica. Il prossimo passo, l'abbiamo detto tutti, è la manovra finanziaria che ci aspetta, quella che oggi è al vaglio del Consiglio dei ministri. È una manovra finanziaria importante che forse, per quel che ho detto, si poteva anche tenere su volumi più bassi. Forse la cifra di cui oggi si parla, pari a 25-27 miliardi,

non possiamo limitarci a misure tampone: dobbiamo impegnarci in riforme strutturali. In questi due anni qualche riforma strutturale il Governo l'ha portata avanti. Voglio citare la più importante, che pure dovrà avere

che il Capo dello Stato in questo momento ci richiama al senso di responsabilità di tutte le forze politiche - certo il dibattito è acceso

sinteticità e stringatezza, è tuttavia un dibattito molto significativo e importante, dato il momento che si sta vivendo. Non mi soffermerò sulle questioni più strettamente tecniche del provvedimento di cui abbiamo avuto modo di discutere in Commissione, in particolare sul fatto che che queste emissioni, per la loro modalità, non creano problemi di sovraesposizione, di offerta eccessiva dei titoli di Stato, perché tutto sommato è una quantità contenuta, con un tiraggio che sarà scalettato nei prossimi anni. Tra l'altro, queste emissioni consentono, nel differenziale tra i tassi attivi e passivi, di avere una remunerazione, da una parte sufficiente per l'esposizione italiana, dall'altra tale da indurre il Paese destinatario, cioè la Grecia, ad adottare comportamenti virtuosi per poter ripagare

superato il primo periodo nel quale, per dirla con Henry Kissinger, l'Europa non aveva un unico numero telefonico, l'Europa è riuscita a trovare la strada della solidarietà

questa volta un po' più solo davanti a se stesso, con la necessità di provvedere a far sì che venissero rimossi quei motivi di difficoltà che in sostanza la crisi greca aveva mostrato in tutta la loro drammatica evidenza, più che altro possono farsi risalire alla scarsa competitività del sistema europeo e alle difficoltà delle finanze pubbliche complessive dei Paesi europei. non è un approccio consolatorio, ma è chiaro che il nostro Paese si trova in una situazione di finanza pubblica non particolarmente rischiosa, perché i suoi fondamentali sono tutto sommato positivi. È vero che il livello del debito è alto, ma il livello del deficit è nettamente inferiore rispetto a quello dei più importanti Paesi europei

operi una serie di riforme, queste sì di carattere sostanziale e strutturale, in modo da far sì che, finita la crisi, il nostro Paese possa presentarsi, per così dire, con le tasche alleggerite dai molti sassi che aveva prima e più pronto a correre quando ci sarà la possibilità di una ripresa internazionale. Sotto questo profilo, le misure che il Consiglio dei ministri adotterà nella giornata odierna complessivamente operano delle sostanziali riforme strutturali nei principali comparti di spesa del nostro Paese, a iniziare dal pubblico impiego, dalla sanità, dai rapporti con gli enti locali, dalla fiscalità. In questo senso, smentiscono l'approccio più cauto che nel passato aveva indotto a evitare di adottare riforme strutturali in periodi di crisi. Questa è una crisi tale che invece pone un obiettivo diverso, quello appunto di cambiare la forma del nostro Paese, di cambiare la la latitudine dell'intervento pubblico, in modo da modernizzare sostanzialmente i meccanismi di entrata e di spesa di questo Paese, che per troppi anni avevano seguito un *trend* tralaticio.

signora Presidente. Sto per concludere. Dicevo che questa è una delle crisi che si stanno susseguendo a partire dalla fine del 2007. Tutti i nodi stanno venendo al pettine. Prima abbiamo avuto una crisi finanziaria, poi una crisi delle finanze pubbliche degli Stati. Vedremo quale sarà l'evoluzione, ma rispetto a questo scenario, difficile e molto in movimento, non si può far altro, ognuno per ciò che attiene alla propria responsabilità, che comportarsi nel modo più prudente possibile e cercare di disinnescare quelle mine che possono portare a danni maggiori nel futuro. Questo è l'approccio con il quale ci siamo mossi, un approccio di estrema prudenza, che consente anche di valutare con preoccupazione, da una parte, ma con legittime aspettative, dall'altra, l'evoluzione dell'euro e dell'Unione europea, perché su questo condivido ciò che è emerso nel dibattito - la crisi ha mostrato una certa limitatezza degli strumenti a disposizione dell'Unione europea, perché il solo strumento monetario è inefficace per poter affrontare le condizioni economiche attuali e anche una seria concorrenza con i Paesi e con le realtà geopolitiche più evolute. Quindi, se l'Europa riuscirà a cogliere da questa occasione lo stimolo per fare un passo avanti verso il consolidarsi di un più stretto rapporto, sia finanziario sia economico sia, soprattutto, politico, credo che qualche effetto positivo questa crisi lo potrà aver avuto. Concludo, signora Presidente, per per rappresentare a questo ramo del Parlamento che le misure che verranno adottate oggi (sulle quali ovviamente ci sarà il massimo dibattito possibile in Parlamento e nel Paese) vorrebbero, nell'intento del Governo, unificare, in una sorta di concordia nazionale davanti alle difficoltà del momento, tutte le parti politiche affinché si possa realmente far fronte alle difficoltà soprattutto delle componenti più deboli del Paese e superare, in un insieme concorde e basato su una forte volontà fattiva, le difficoltà che abbiamo di fronte oggi, che non sono di per sé assolutamente insuperabili.

potrebbero dare dei comandi decisamente troppo forti al Governo. In alcuni casi è meglio avere un approccio più morbido, soprattutto per quanto riguarda i rapporti internazionali. Per questo motivo, apprezzandone lo spirito, se i presentatori sono d'accordo, sono disposto ad accoglierli

raccomandazione perché, pur con tutto il senso di responsabilità che l'Italia dei Valori ha, sono due anni che ci stiamo raccomandando al Governo e non possiamo più proseguire oltre.

Signora Presidente, la Grecia e l'Italia: da un lato, le manifestazioni in piazza ad Atene fino ai morti, fino alla tragedia; dall'altro, la protesta operaia a Milano, a Termini Imerese, in Sardegna e in tanti altri luoghi, protesta che inventa anche forme di lotta clamorose, dettate dalla paura di fronte al rischio della povertà o all'assenza della politica. Raccontano entrambe di una crisi seria, grave, emergenziale, al di là delle tante chiacchiere di chi un giorno la vede superata e un altro giorno la vede così così. Anche abbiamo percepito da parte del Governo solo un proclama di intenti tardivo, di regole da consegnare al sistema finanziario, come se la crisi non fosse assieme crisi di un sistema finanziario e di un modello di coesione sociale. ci ha rassicurato - il sottosegretario Letta per spiegare al Governo che la situazione economica è serissima. Sono sue le parole «una serie di sacrifici molto pesanti, molto duri (...) per salvare il nostro Paese dal rischio Grecia. Capiamolo così e ci capiamo tutti». Sono queste le sue parole. Noi dell'Italia dei Valori e gli italiani l'avevamo capito e detto da tempo. E da qui dobbiamo partire se vogliamo capire sino in fondo una situazione folle come quella che sta vivendo la Grecia, dove succede che a dettare le condizioni dell'assetto sociale siano le banche e non la politica. Da una parte, i sedici Paesi della zona euro che hanno adottato la stessa moneta, ma non riescono a dotarsi di una politica economica comune; dall'altra, il mercato e la speculazione, le grandi banche d'affari, gli *hedge* *fund*, che prendono di mira i titoli di Stato dei Paesi più in difficoltà sul fronte dei conti pubblici (e le armi più utilizzate sono la vendita allo scoperto, una sorta di scommessa sulla perdita e sulla sconfitta di un Paese, di una comunità). Da qui dobbiamo partire per capire che questa crisi, che chiamiamo finanziaria, è a tutti gli effetti una crisi reale. Quello che è successo è stato anche, ma non solo, un eccesso di debito che è andato su spese inutili e sui consumi, e ora la finanza chiede i soldi indietro. In Italia, quindi, non siamo affatto oltre la crisi, come ci si diceva sino a pochi giorni fa. Per l'occupazione siamo nella fase peggiore. Ma la crisi serve al Governo e ad alcuni settori per dettare nuove relazioni sociali. Si parte con l'accordo separato sul sistema contrattuale, si continua con il collegato sul lavoro, si mette in mezzo la riduzione delle tutele sul lavoro e l'aumento della precarizzazione. Tra novembre 2008 e aprile 2010 sono stati emanati ben sette decreti‑legge di pertinenza economica. In questi giorni si parla molto, dopo l'intervento del presidente Napolitano, di equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento, e i decreti-legge spostano, naturalmente, l'equilibrio in una direzione pilotata dal Governo. Ma qui c'è qualcosa di più preoccupante e più grave: la frammentazione della politica di bilancio, con una perdita di trasparenza delle scelte e dei risultati delle stesse sui conti pubblici che rende molto più difficile qualsiasi discussione informata sulla finanza pubblica. Mentre servivano riforme credibili per ritornare alla crescita, mentre servivano manovre che non facessero aumentare la spesa e il deficit pubblico, ma che finanziassero gli investimenti, il Governo ha propinato al Paese un insieme disorganico di micromisure e di interventi parziali, dal *bonus* temporaneo alle famiglie povere ai numerosi microincentivi che, disperdendosi in mille rivoli, sembrano più adatti a massimizzare, sul piano elettorale, il numero dei potenziali beneficiari che a fronteggiare davvero la difficile situazione economica.

La prima è che il decreto-legge di aiuti alla Grecia, e con esso il difficile e complesso piano di salvataggio, non nasce dai 50 minuti di telefonata di Silvio Berlusconi impiegati per convincere Angela Merkel a dare il via libera, come racconta Bruno Vespa nel suo ultimo libro. In questo, Berlusconi ha saputo trasformare anche la tragedia greca in una caricatura della democrazia. La Germania, con il ricostituito asse franco-tedesco, con le sue banche e la sua economia, ha più interesse di tutti a salvaguardare i mercati finanziari e a richiedere più coordinamento e, soprattutto, più riforme strutturali, per eliminare l'eccesso di sprechi nella spesa pubblica. La seconda certezza: nella manovra che il Governo sta varando non è, come sostiene Tremonti, che ora e soltanto ora i tempi delle correzione sono imposti dalla crisi. Lo erano già da prima! Da tempo abbiamo chiesto di definire il perimetro dell'aggiustamento dei conti pubblici fissando alcuni paletti. Il Governo ha risposto con condoni e con lo scudo fiscale, le cui entrate tra l'altro non verrebbero neppure contabilizzate come parte dell'aggiustamento. Da tempo abbiamo chiesto che gli effetti delle misure adottate non fossero sovrastimati: non possiamo permettercelo dopo i trucchi contabili della Grecia. Abbiamo chiesto che il Governo desse un segnale forte nel contrasto all'evasione, e sin qui il Governo non ha voluto farlo, teorizzando di non voler appesantire con la burocrazia le imprese durante la crisi. Abbiamo chiesto che non ci fossero interventi volti a fare cassa nell'immediato, aumentando poi gli impegni di spesa futuri, come ad esempio la prospettata chiusura delle finestre per le pensioni di anzianità, che può servire a ridurre temporaneamente le spese, per aumentare quelle future, con il risultato di risparmi strutturali residui. Da tempo abbiamo chiesto di non procedere in modo indiscriminato con tagli lineari e uguali per tutti. Solo adesso ci si accorge che ci vogliono 24 miliardi nei prossimi due anni, più di quanto ogni anno spendiamo per difesa e istruzione universitaria messi insieme. Il ministro Tremonti, nella sua nota trasmessa e letta alla Camera dei deputati sullo stato della Grecia, ci ha ricordato che «è sbagliato guardare con occhio nazionale alle cose europee». E ce lo ha ricordato mentre alternava in questi due anni, nella sua politica economica, lo strabismo alla cecità. Ricordiamo tutti la finanziaria del 2008, approvata dopo nove minuti e mezzo. Conteneva la stretta fiscale per i banchieri e i petrolieri. Quando la situazione delle banche è precipitata dopo il fallimento della Lehman Brothers, Tremonti si è vantato di aver previsto tutto anticipando la presentazione della finanziaria. In realtà poi i dati sono lì a dimostrare gli effetti nulli della Robin *tax*.

ha giudicato ogni norma proveniente dall'Europa come lacci e lacciuoli soltanto in grado di frenare la libera iniziativa. È sua l'affermazione nel 2008 secondo cui «bisogna evitare di rompere le scatole alla gente con un eccesso di regole», e oggi viene a dirci che se il male è stata l'assenza di regole, la cura può essere solo nella costruzione di regole. in queste settimane ad aver notato che il Governo, dopo aver abolito e demonizzato tutte le misure antievasione introdotte dal Governo Prodi, ne sta, gradualmente e purtroppo tardivamente, recuperando alcune, dopo che i buoi sono scappati dalla stalla. L'Italia non è la Grecia, si è detto ed è vero: a differenza della Grecia, il nostro è un grande Paese industriale. Tuttavia i livelli di illegalità e corruzione nei due Paesi risultano molto simili. E su questo è necessario che ci sia una riflessione da parte di tutti, soprattutto nel nostro Paese, dove la principale causa di ingiustizia sociale resta ancora la sperequazione fiscale. Diciamola così, in poche parole, su questo decreto-legge, mettiamola in questo modo: una spregiudicata attività internazionale di speculatori dell'alta finanza decide da New York, Lussemburgo o Shanghai una razzia ai danni di alcune dissestate Nazioni d'Europa. E i governanti delle nostre Nazioni cosa fanno? Per ergere una barriera finanziaria a difesa della loro gente non trovano di meglio che salassare ulteriormente i già vessati salari del pubblico impiego e dei pensionati. Questo è l'aspetto che deve farci riflettere e preoccupare. signora Presidente, concludo. Se gran parte delle misure, mezze annunciate e mezze smentite dal Governo, si tradurrà in fatti nella prossima manovra economica, il Governo non avrà più titolo per dire di «non aver messo le mani nelle tasche dei cittadini». È l'ultima menzogna di questo Governo. Per queste ragioni, il voto dell'Italia dei Valori sarà contrario.

il nostro Gruppo parlamentare ha deciso di votare a favore del decreto sugli aiuti alla Grecia. Abbiamo deciso di sostenere questa misura del Governo perché riteniamo che sarebbe da irresponsabili fare altrimenti e, come è noto, la responsabilità è da sempre una delle nostre principali cifre distintive. Responsabilità, sia ben chiaro, in primo luogo verso i cittadini italiani risparmiatori, che non possono essere abbandonati a se stessi in frangenti drammatici come quelli che stiamo vivendo; responsabilità che significa infondere nei cittadini la giusta fiducia, far sentire loro che non sono soli ma che le istituzioni sono attive nel tutelare i loro interessi; responsabilità verso gli italiani, perché il provvedimento che votiamo oggi, che prevede lo stanziamento di aiuti alla Grecia per un impegno massimo di quasi 15 miliardi di euro è, in realtà, un decreto che ci riguarda tutti, ci riguarda tutti, e molto da vicino. I prestiti che oggi accordiamo alla Grecia non vanno solo a sostegno del Paese ellenico; sono una misura per sostenere e rafforzare l'euro, che in queste settimane è stato messo sotto attacco dalla speculazione internazionale. E se, dunque, salvare la Grecia significa rafforzare l'euro, approvare oggi queste misure equivale a rendere più forte e più sicura l'intera area economica e monetaria di cui l'Italia è socia fondatrice e parte integrante. Salvare oggi la Grecia significa creare le condizioni per cui non si sia costretti a dover salvare l'Italia. Questa, infatti, cari colleghi, dev'essere un'occasione per rafforzare l'Unione europea e non per scioglierla; per fare ciò è necessario - e noi in questo senso abbiamo votato anche alcuni ordini del giorno presentati dal collega Lannutti - anche rivedere un sistema di regole che fa affidamento sulle agenzie di *rating* che sono obiettivamente inaffidabili come rischiano di determinare, il *default* della Grecia rispetto alla valutazione dei titoli di Stato dalla stessa emessi con una disinvoltura che nessuno ormai può più permettersi. Certo, Certo, signora Presidente, alcuni problemi relativi al rifinanziamento del debito pubblico italiano possono esservi ed incidere anche in ordine alla concessione dei prestiti alla Grecia. Un Paese come il nostro, infatti, vincolato da un enorme debito pubblico, potrebbe essere esposto ad una crisi fiscale nella misura in cui sarà costretto a ricorrere ai mercati per il rifinanziamento del suo debito. Tutto ciò è ovviamente legato a quanto debito pubblico scadrà nei prossimi mesi e, a seguire anche, alla cosiddetta scadenza media del nostro debito. Se il nostro debito è a lunga scadenza, la quantità da rifinanziare in un dato tempo è piccola ed il costo sopportabile, ma se il debito è a breve termine ed è quindi elevato lo *stock* da rifinanziare il rischio di crisi fiscale è forte. E di certo gli aiuti alla Grecia nel breve periodo aggravano l'ammontare del debito pubblico, in quanto il Tesoro utilizzerà le aste titoli già in programma ampliandone l'offerta. È quindi evidente che noi dobbiamo sostenere questo ampliamento delle offerte dei titoli del debito pubblico. E l'unico sostegno possibile è una sostanziale inversione di rotta nella nostra politica economica. maggior rigore nella gestione dei conti pubblici per rafforzare la fiducia dei mercati e rendere quindi sicuramente appetibili anche queste nuove emissioni. Voglio ricordare a tutti che, per quanto la situazione odierna della Grecia possa sembrare difficile e il suo salvataggio si stia rivelando molto oneroso, se domani l'Italia si dovesse trovare in una situazione analoga, salvarla sarebbe molto più complesso e costerebbe molto di più di quanto oggi siamo impegnati a stanziare per la Grecia, anche e soprattutto in relazione alle dimensioni del nostro debito: un debito che - è bene lo teniamo tutti sempre a mente - viaggia nell'ordine del 115 per cento del nostro prodotto interno lordo. Noi dunque agiamo oggi con senso di responsabilità, valutando con spirito critico e senza pregiudizi l'operato dì un Governo che ha saputo allinearsi alle decisioni europee, evitando la tentazione di smarcarsi o di cercare un compromesso al ribasso. Da convinti europeisti quali siamo chiediamo anche a tutti i nostri partner europei, qui ed oggi - ma faremo altrettanto, mi auguro, anche nelle sedi istituzionali comunitarie - di agire con la stessa energia e con la stessa convinzione con cui oggi l'Italia, con il suo Parlamento, sta reagendo, assicurando un pieno sostegno al piano di aiuti europeo. Oggi, come detto, sosteniamo il pacchetto di aiuti proposto dal Governo, non solo perché nel breve e nel lungo periodo potrà convenirci, stando al differenziale tra gli interessi pagati tra gli interessi pagati dalla Grecia sul prestito e gli interessi che paghiamo a chi sottoscrive questa emissione di titoli, ma soprattutto perché riteniamo opportuno avviare con questo provvedimento una manovra più complessiva che riguarda anche il risanamento della nostra economia. Sappiamo bene che questa misura, approvata nell'emergenza e nell'urgenza di una situazione che si stava facendo esplosiva anche sul piano sociale, e che rischiava di avere ricadute a cascata difficilmente prevedibili anche sull'Italia, è appunto di carattere emergenziale: una rete posta per evitare la frana, ma che non risolve le problematiche strutturali che quella frana ha generato, non incide in maniera decisiva sulle cause che ci hanno portato nella situazione in cui oggi ci troviamo

Quello che dobbiamo allora avere a mente anche per i provvedimenti che saremo chiamati ad esaminare in quest'Aula nelle prossime settimane è che l'attuale situazione greca è stata frutto di una serie di concause ma trova però il suo fulcro in un elemento essenziale: la mancanza di rigore nei conti pubblici. Le vicende di oggi devono allora servirci come monito a non dimenticare mai che questa deve essere la regola - abbondantemente tralasciata anche da questo Governo che ci mette al riparo da problemi come quelli che si stanno vivendo in questo Paese. Nuove e più incisive misure dovranno dunque essere messe a punto ed approvate, e credo lo saranno a breve, come apprendiamo anche dalle notizie di stampa di oggi. Ed è bene che ciò avvenga, sicché ci aspettiamo con serenità, quando avremo modo di discutere questa manovra economica, il Ministro dell'economia venga in Parlamento e ci dica con grande chiarezza qual è la situazione dei nostri conti pubblici, quale l'entità della manovra, quali sono le misure concrete con cui a quella manovra si intende dar vita. Quando vedremo questi dati, i numeri, le coperture, i saldi e tutto quanto necessario, daremo la nostra valutazione e, ancora una volta, sarà una valutazione scevra da pregiudizi, che consentirà anche a noi, nonostante siamo un Gruppo parlamentare di opposizione, di assumerci la responsabilità di concorrere con spirito costruttivo alla definizione di provvedimenti che facciano bene al nostro Paese. Aspettiamo quindi di studiare la manovra nei suoi particolari prima di pronunciarci, anche se alcune cose credo che possiamo dirle. alcune cose credo che possiamo dirle. La prima è che non si può accettare che il peso principale di questa manovra possa gravare sulle spalle delle famiglie italiane, dei giovani, di coloro che restano ai margini del mercato del lavoro, delle fasce sociali più deboli. Né possiamo ritenere che questa crisi diventi una nuova occasione di frattura sociale e generazionale, anche perché le nostre famiglie, le famiglie italiane, sono state già duramente colpite dalla crisi economica internazionale, che fa sentire da più di due anni i suoi morsi. La disoccupazione ha rialzato la testa dopo anni di progressiva diminuzione e, almeno per il momento, non dà segnali di ripiego. È pur vero che alcuni segnali, ad esempio quelli riguardanti la produzione industriale, possono sembrare incoraggianti. Ma si tratta ancora di segnali flebili, isolati, che che comunque da soli non sono in grado di darci un quadro obiettivamente ottimistico. Servono misure incisive, soprattutto servono misure strutturali, che ci facciano finalmente uscire dalla logica dell'emergenza con cui fino ad oggi è stata affrontata la maggior parte dei problemi di ordine economico del nostro Paese. Servono misure che, mettendo insieme equità e lungimiranza, permettano un'inversione di tendenza del nostro debito pubblico, da riportare possibilmente sotto il 100 per cento del PIL entro la fine di questa legislatura, consentano un graduale rientro del deficit entro i parametri del patto di stabilità, come concordato con la Commissione europea, e allo stesso tempo pongano le basi per una ripresa solida, robusta e duratura della nostra economia nazionale. Misure, dunque, che sappiano coniugare tenuta dei conti pubblici e rilancio dell'economia. Sappiamo che non è semplice, anche in considerazione dei margini di manovra della politica fiscale che in Italia sono certamente angusti, ma è il momento di agire con decisione, rinunziando alla tentazione dei meri *maquillage* contabili che altre volte abbiamo visto, tagliando le spese inutili in modo strutturale, magari seguendo l'esempio di Germania e Francia, che stanno approvando leggi costituzionali che impongono ai Governi la promozione di piani di ridimensionamento del debito pubblico con obiettivi vincolanti. Oggi, signora Presidente, diciamo sì al decreto di aiuti alla Grecia, invitando l'Esecutivo a vigilare sull'impatto che questi nuovi prestiti potranno avere sui conti italiani, ma riconoscendo che in questa circostanza il Governo ha operato in maniera tempestiva. Siamo pronti ad assicurare uguale sostegno a misure che, con quelle stesse caratteristiche, vadano ad incidere sui conti pubblici del nostro Paese e a quelle misure siamo pronti a dare il nostro contributo nelle Aule parlamentari, al fine di renderle efficaci. Senza pregiudizi, ma senza firmare cambiali in bianco.

Si sa che, nel lungo periodo, un'unione monetaria senza un'unione politica non può esistere: ora si tratta di capire se il lungo periodo è lontano, oppure drammaticamente vicino, e questo ancora oggi non lo sappiamo. Si sa anche che per avere una moneta unica servono diverse condizioni, ed in particolare due: un'area economica omogenea (e l'area economica omogenea non c'è) ed una mobilità dei fattori produttivi, in particolare del fattore lavoro, sufficientemente elevata. Ma se negli Stati Uniti è normale che un texano si trasferisca a Washington o in Alaska, in in Europa semmai ci sono dei trasferimenti dal Sud Europa verso il Nord Europa: è difficile che un finlandese si trasferisca in Italia, in Grecia o in Spagna. Ci sono quindi dei problemi abbastanza seri, complicati dall'allargamento. Si sa che la Lega è stata critica sull'allargamento, senza valutarlo fino in fondo, su tutti i suoi aspetti, anche per considerazioni ovvie e banali. Non so quanti colleghi in quest'Aula si ricordano qual è la capitale dell'Estonia o della Lituania o quale lingua parlano in quei Paesi, e meno e meno male che non parliamo più di Turchia, per il momento. La situazione è davvero complicata, ma l'euro è la nostra moneta ed è nostro dovere oggi difenderla, questo è un dato di fatto. Come più colleghi hanno correttamente fatto rilevare, la speculazione non è la radice, ma è l'effetto di un fenomeno. Come diceva Einaudi, lo speculatore è come il coniglio: è veloce ma è un fifone,

allora assolutamente logico che i mercati siano scettici con la Grecia e la Spagna, che hanno un grande debito pubblico ed una disoccupazione al 20 per cento: è chiaro che qualcuno si ponga la questione se ce la faranno a ripagare i debiti.

Siamo messi benissimo come aziende (siamo infatti sotto la media) ma, a livello di debito pubblico, siamo i peggiori di tutti, e ci supera purtroppo solo la Grecia: abbiamo quindi un problema serio, un problema debito, e lo sappiamo tutti.

sul settore pubblico, sul debito e sul peso del settore pubblico, per cui occorre ridurre il Leviatano: dobbiamo ridurre il peso dello Stato, non si può fare altro, e la manovra non può che andare in questa direzione. Inoltre - e questa è una peculiarità tutta italiana - è enorme la disomogeneità all'interno del nostro Paese. Le differenze tra Nord e Sud in tutte le classifiche sono molto molto rilevanti: abbiamo mezzo Paese, dal Nord fino alla Toscana, con i fondamentali della Germania, e mezzo Paese, purtroppo, con i fondamentali di Grecia e di Spagna. Questo è il dato di fatto e questo è, insieme alla riduzione del peso dello Stato, l'altro problema che dobbiamo

È assolutamente chiaro, per noi della Lega Nord, che questa è l'unica riforma strutturale possibile, prima che sia troppo tardi, e speriamo che anche gli altri colleghi si rendano conto di qual è veramente la situazione. *(Applausi

Siamo convinti che in questo caso il Governo abbia salvaguardato l'interesse nazionale. Non si trattava, infatti, di una solidarietà a favore di uno Stato in difficoltà. Si è trattato e si tratta di svolgere un'azione efficace in difesa dell'euro, della forza di una moneta unica che costituisce un ancoraggio essenziale per il nostro Paese. Abbiamo anche apprezzato la scelta di campo, questa volta senza equivoci, a favore di più Europa, superando un passato che era stato caratterizzato da timidezze e dalla tentazione del populismo, accreditando nell'opinione pubblica l'idea che l'Europa fosse un ostacolo e un'occasione di difficoltà e non piuttosto una risorsa. Del resto, la crisi dimostra che la grande scelta dell'euro, sostenuta da una lungimirante visione politica di leader di levatura europea, e la grande scelta lungimirante di Prodi e di Ciampi di fare dell'Italia

richiede che la moneta unica si accompagni ad una maggiore cooperazione fiscale dal lato della spesa e dal lato del prelievo, altrimenti, questo progetto, questa realtà entrerebbero in una difficoltà insuperabile. Regole troppo diverse, competizioni fiscali al ribasso rendono meno competitivo il continente europeo. Lo abbiamo sostenuto in passato, lo sosteniamo oggi. Ci fa piacere che il Governo oggi se ne sia reso conto, ma ora occorre procedere con coraggio. Le difficoltà del Parlamento europeo di approvare un atto di indirizzo dei Governi di fronte alla crisi dimostrano che occorre agire con determinazione per questo passo ulteriore, che non è affatto scontato. La lezione della Grecia serve anche per noi. Se un Paese non cresce, se l'avanzo primario viene azzerato, se il debito continua a crescere, è chiaro che questo debito non è più sostenibile. In questo caso, è vero, non c'entra nulla la speculazione internazionale, anche se vorrei dire al senatore Grillo che la speculazione internazionale esiste, e non si chiama "mercato" un ambito senza regole. L'attacco che l'euro sta subendo non è figlio del funzionamento del mercato, ma è figlio di decisioni di ben individuati gruppi finanziari. c'entra nel fatto della Grecia che banche stressate hanno investito troppo in titoli ad alto rendimento, ma troppo rischiosi; semmai c'entra il fatto che la scelta opaca dei Governi porta alla situazione - come ricordava la presidente Bonino - che in Europa si possono truccare i conti da parte dello Stato. Attenzione, la Grecia è un *memento* anche per noi. L'Italia ha, per fortuna nostra, dei fondamentali molto diversi da quelli della Grecia, come base produttiva, come specializzazione produttiva, come bilancia commerciale, come peso della componente pubblica; abbiamo un dato in comune: il debito pubblico della Grecia è il 115,1 per cento del PIL. A legislazione vigente, l'Italia sarebbe, a fine 2010, al 118,4 la drastica manovra che il Governo annuncia non ha nulla a che fare con la Grecia: ha a che fare con i nostri ritardi, con le nostre insufficienze, anche con il tempo perso da questo Governo. Ricordo che l'ultimo bilancio firmato dal Governo di centrosinistra aveva un debito al 103,5 per cento del PIL; dopo due anni di cura del Governo di centrodestra, il debito è salito a 115,8 per cento. Non basta la solita storia del denominatore e del numeratore: il PIL è sceso, ma le spese sono enormemente aumentate. In due anni, 51 miliardi di spesa pubblica in più, il doppio della manovra che ora richiedete al Paese, e che si sarebbe evitata se questi 51 miliardi fossero stati posti sotto controllo. Per questo, guardiamo con profonda preoccupazione all'annuncio della manovra presentata dal Governo. Ne discuteremo naturalmente nei prossimi giorni, ma è chiaro ed evidente che in questa manovra resta la costante che ha caratterizzato la vostra azione: la parola "riforme" non esiste. Non solo non esiste la parola, ma non esiste neanche l'ambizione. Ancora una volta la manovra su cosa si regge, per quello che possiamo capire? Su un condono fiscale, sotto forma di un mega condono edilizio, un taglio ulteriore al sistema delle autonomie locali. Senatore Garavaglia, siamo con lei nel sostenere che il federalismo, se se ben attuato, è una strada essenziale per il futuro del Paese. Questo federalismo, però, non può essere una promessa per il futuro. La realtà amara è che oggi centralizzate ancora di più e fate pagare al sistema delle autonomie l'incapacità dell'azione di controllo della spesa centralistica. Portate più Stato e più inefficienza della spesa, e questo è veramente inaccettabile. I tagli che fate alle Regioni e ai Comuni produrranno questo. Le Regioni taglieranno quella parte di risorse che trasferiscono ai Comuni e questi saranno l'unico terminale. Ciò vuol dire distruggere il *welfare* di sostegno alle famiglie. Vuol dire distruggere quella capacità di stazioni appaltanti diffuse che sostengono il sistema della piccola e media impresa nel settore delle costruzioni, e non solo. Poi c'è la ricetta Certo, la spesa pubblica deve essere resa più efficiente, ma dovete intervenire nei meccanismi di formazione della spesa. Esistono risultati Esistono risultati davvero importanti della Commissione per la spesa pubblica, presieduta dal professore Gilberto Muraro, che voi avete chiuso. Basterebbe esaminarli. C'è un manuale di risparmi possibili. Perché non li attuate? Se non introducete sul serio un criterio di valorizzazione del merito dell'efficienza nella pubblica amministrazione, come pensate di riuscire a controllare *ex post*? L'avete già fatto nel 2008 e nel 2009 e i risultati non ci sono stati. Ancora una manovra fatta di *una tantum*. l'insegnamento della Grecia. Far finta di niente è il modo peggiore di risolvere i problemi. Lo avete fatto per due anni. Nell'interesse del Paese vi chiediamo di non farlo ancora nel futuro. Usate parole di verità nei confronti dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica è più matura di quanto voi possiate pensare. È in grado di comprendere il segno di sacrifici, purché siano distribuiti in modo equo: la manovra non registra un'equità di opposizione di sacrifici ai vari gruppi sociali del Paese. E purché questi sacrifici siano utili: la cosa peggiore è chiedere sacrifici inutili, perché prendete solo un po' di tempo e, tra due anni, il Paese starà in condizioni peggiori di quelle attuali.

il Presidente del Senato e il Governo abbiano dato prova dell'assoluta responsabilità istituzionale, peraltro una responsabilità sollecitata da tutto il Parlamento. Oggi, al di là delle urla e degli strepiti che di solito circolano in giro per la Nazione, si scrive una bella pagina parlamentare e istituzionale. Detto questo, vorrei ricordare a tutti come si giunge al provvedimento in esame, la cui breve ricostruzione è essenziale per comprendere in fondo il convinto voto favorevole che esprime il Gruppo del Popolo della Libertà. Desidero ricordare a tutti che, nel corso della grave crisi finanziaria del biennio scorso, grazie ad un'oculata attenzione e ad una oculata politica del Governo, del Governo, lo Stato italiano è stato quello che ha avuto minori uscite pubbliche per affrontare la crisi. tutti gli altri Stati hanno dovuto produrre misure di gran lunga più incisive e dunque hanno allargato la spesa pubblica in maniera considerevolmente superiore a quanto

Quindi, la critica che ci viene mossa è ingiusta. L'aumento del debito pubblico italiano in questi anni è stato considerevolmente inferiore a quello degli altri Paesi. conto di una condizione di partenza molto più onerosa, è evidente che ciò impone misure altrettanto importanti, cosa di cui il Governo ha piena coscienza.

sul PIL tra i Paesi occidentali. Ciò significa che in questo periodo, nonostante il gravoso onere del debito, è stato possibile attuare un significativa correzione dei conti che ci ha portato ad una situazione in cui il nostro deficit più facilmente di altri può rientrare nei parametri di Maastricht.

assolutamente negare; successi che sono stati conseguiti grazie all'azione del Governo. Ma vi è di più. Voglio ricordare la parte attiva, direi rilevante e riconosciutaci da tutti, che il Governo ha avuto nella stesura di questi provvedimenti.

nella definizione dei provvedimenti che hanno posto riparo alla gravissima crisi di finanza pubblica dei giorni scorsi.

dell'Unione europea per fronteggiare la crisi di finanza pubblica, dall'altro, che riteneva necessario un incisivo passo avanti nella costruzione dell'Unione europea politica per poter consolidare l'euro. L'Italia è da tempo che individua in una moneta senza Stato uno dei problemi più gravi che oggi l'euro vive,

Colleghi, vi chiedo la cortesia di consentire al senatore Azzollini di concludere la sua dichiarazione di voto in un'atmosfera più consona.

Stato per Stato e nei tempi più brevi possibili, per tagliare le unghie alla speculazione nei confronti dell'euro. Questo è quanto ci stiamo apprestando a fare con la manovra. Certo, sono state fatte alcune considerazioni, secondo me, anche importanti e che hanno una certa fondatezza, cioè la necessità di inserire i provvedimenti urgenti e necessari in un quadro di provvedimenti che incida anche sul medio e lungo periodo.

Ai colleghi che hanno detto che è aumentato il debito pubblico, ricordo che certamente è aumentato, ma in misura minore rispetto a tutti gli altri Stati occidentali. Oggi il problema che avremo di fronte è però il seguente. Com'è noto, il debito e il deficit e si misurano con un'altra grandezza, quella del prodotto, quindi della crescita. È evidente c'è bisogno che l'Italia ritrovi competitività per il suo sistema industriale, che l'Italia ricominci a riequilibrare la bilancia commerciale, che l'Italia torni ad essere la sesta potenza del mondo, anche sul piano della sua industria, ma non possiamo non ricordare che soltanto una finanza pubblica pienamente sotto controllo può favorire lo sviluppo dell'economia. dell'economia. Non abbiamo ricette precostituite. Sarebbe facile se ci fossero. Ogni giorno l'azione dei Governi deve tenere conto dell'insieme delle situazioni che si presentano loro dinanzi e dei grandissimi movimenti di capitale che di giorno in giorno si spostano spostano dall'uno all'altro investimento, con dimensioni inaudite: inaudite, nel senso che mai erano state affrontate prima. Per questo, il Popolo della Libertà

dal Governo italiano nel corso di questi due anni di gravissima crisi industriale e di finanza pubblica. Oggi abbiamo di fronte le sfide del futuro. Ciò che abbiamo fatto mi sembra un'ottima premessa per far bene in seguito. Naturalmente la maggioranza dovrà monitorare tutto quello che verrà fatto, ma lo faremo sempre con questo puntuale spirito costruttivo. Un'ultima cosa. Il Presidente della Repubblica ha richiamato in questi giorni che i sacrifici devono essere equi. Non vi è dubbio che il concetto di equità è da questa maggioranza e da questo Governo da tempo espresso, e noi riteniamo che tradurrà in provvedimenti che alla necessità del rigore coniugheranno la necessità dell'equità, così da avere una manovra equilibrata nel suo complesso. Per questo, signora Presidente, il Gruppo parlamentare del Senato del Popolo della Libertà voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

accelerata interrogazione in istantanea per un incontro che avverrà domani tra un'importante delegazione dei lavoratori Eutelia e la prefettura, dopo un assai difficoltoso incontro avvenuto con l'assessore regionale e con il Governo, che non si è però presentato. Si tratta di 300 lavoratori a Torino e Ivrea

e ha avuto anche momenti di durezza: una formale e breve occupazione dell'assessorato da parte di una delegazione. Domani si terrà finalmente un incontro in prefettura e mi auguro che il Governo sarà presente per assumersi quegli impegni presi nel novembre del 2009 e purtroppo disattesi, con gravissime situazioni di disagio economico per centinaia di lavoratori. **Per

al Governo di informare il Senato in merito alle circolari che stanno arrivando nelle scuole italiane ai dirigenti scolastici e persino agli insegnanti. circolari intimidatorie aventi lo scopo di impedire loro di informare i genitori della reale situazione finanziaria e di personale delle scuole; per informarli, insomma, di quello che li aspetta il prossimo anno. La consapevolezza della situazione arriva alla coscienza dei genitori solo adesso - il ministro Gelmini dovrebbe sapere bene proprio perché gli stessi soggetti (insegnanti e dirigenti scolastici) l'anno scorso hanno tamponato finché hanno potuto. Ma adesso, come si suol dire, siamo alla canna del gas:

che poi abbiamo visto anche negli anni Cinquanta in alcune fabbriche italiane. Trovo ciò molto grave, e vorrei che lei chiedesse al Governo di venire a riferire. Si tratta di fatti gravissimi, che spero non siano riferibili al Ministro, ma a qualche burocrate troppo zelante.

Mentre il Governo vara manovre che vanno a penalizzare solo gli onesti, i lavoratori e i dipendenti statali e che premiano gli evasori e i grandi capitali, nel Lazio stanno chiudendo oltre 200 imprese. Fra queste c'è anche il caso della Nexans, che chiuderà i battenti a fine maggio, causando il licenziamento di 300 lavoratori. È la fine di un'impresa storica del capoluogo pontino, la ex Fulgorcavi, che produce cavi di media e alta tensione, acquistata dalla multinazionale francese quando aveva 1.200 dipendenti, poi ristrutturata, o meglio destrutturata, fino ad arrivare a 300 dipendenti che stanno rischiando il posto. Quanto denunciano gli operai è una precisa volontà, da parte del *management* francese, di non investire né in termini di macchinari né di conoscenza, avendo gli stessi anche rifiutato ordini e commesse per giustificare la chiusura del sito produttivo. Il caso Nexans è solo l'ultimo di una lunga serie di aziende della provincia pontina che vengono dismesse dalle multinazionali per investire altrove. si sono incontrati al tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico i sindacati e l'azienda, che non ha neanche mandato un dirigente, ma solo un impiegato, a dimostrazione dell'alto interesse. Nella riunione è stata ufficializzata la decisione di chiudere e, sebbene si sia arrivati ad una mediazione, ossia il congelamento della trattativa al 1° giugno, giorno del nuovo incontro, sembra molto difficile che ci siano margini di manovra. sarebbe perciò auspicabile che la Presidenza si faccia carico della vicenda per sensibilizzare sia la Presidenza del Consiglio che il Ministero per riuscire ad agire sulle istituzioni francesi e cercare una soluzione che

Grazie,